Comunico all'Assemblea che il senatore Antonio D'Alì ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura - prevista dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione e disciplinata dagli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - per la richiesta di *referendum*, da parte di un quinto dei componenti del Senato della Repubblica, sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», approvato dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione - a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi, dei suoi componenti - nella seduta del 12 aprile 2016, come comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Su proposta del senatore D'Alì, i senatori Vito Claudio Crimi, Loredana De Petris e Gian Marco Centinaio sono stati designati quali delegati a depositare la richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della richiamata legge n. 352 del 1970. Il *quorum* per la presentazione della richiesta di *referendum* è di 65 firme. La richiesta dovrà pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione del predetto comunicato e cioè entro il 15 luglio 2016 (articolo 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352). I fogli per la sottoscrizione della richiesta di *referendum* sono a disposizione degli onorevoli senatori presso la Sala Pannini di Palazzo Madama fino alla conclusione della seduta odierna.

provvederanno all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola: avevo preparato un discorso serio, circostanziato e l'avevo scritto per essere preciso preciso e puntuale davanti al Presidente del Consiglio e al Governo tutto, ma, francamente, mi rendo conto di non farcela. Non ce la faccio a leggere quello che avevo preparato, perché sono arrabbiato. Sono molto arrabbiato

Sono arrabbiato anche perché il signor Presidente del Consiglio, a febbraio del 2014, se ne venne in quest'Aula con una citazione della della canzone di Gigliola Cinquetti «Non ho l'età». A me sembra invece che, in questi mesi di Presidenza del Consiglio, abbia dimostrato di avere ben altro pelo sullo stomaco rispetto a una persona che «non ha l'età». Lo ha dimostrato ampiamente e lo hanno dimostrato molti componenti del suo Governo. Sono arrabbiato, signor Presidente, perché questo Governo ha una tendenza, automatica e continua, a sminuire le cose importanti, a farle passare sotto traccia, a nascondere la polvere sotto al tappeto e il caso di cui parliamo, in questa occasione, che non è soltanto un caso giudiziario, ma è eminentemente e profondamente politico, lo dimostra ancora una volta. È un caso in cui abbiamo visto emendamenti a favore delle *lobby* introdotti a notte fonda alla Camera dei deputati, in maniera agile, da un Ministro per i rapporti con il Parlamento che, essendo giovane come il Presidente del Consiglio, ha mostrato tanta e agilità nell'inserire emendamenti che favorivano le società petrolifere e le società che con quelle lavorano, da dimostrare poi la stessa agilità nel cercare di tirarsene fuori e nel dire che non aveva alcuna responsabilità. Questo non è un comportamento adatto ad un Ministro per i rapporti con il Parlamento. E questo Governo - lo voglio ripetere ancora una volta - sta facendo di tutto per troncare le polemiche, per nascondere le questioni importanti e per riportarle solo ed esclusivamente esclusivamente alla vicenda giudiziaria, sminuendola e definendola roba di poco conto. Bene, la questione giudiziaria non è roba di poco conto, ma vede coinvolto il Governo nella sua completezza,

riconoscere che l'abitudine del Presidente del Consiglio di tenere sotto traccia le questioni importanti nasce certo con lui, almeno per quanto riguarda la Basilicata e le questioni delle*lobby* del petrolio. L'ha inventata il senatore Paolo Romani, allora esponente nel Popolo delle Libertà, che disse, quando era Ministro dello sviluppo economico: «Ma che volete che stiamo facendo con le concessioni ai petrolieri? Faremo sì e no quattro buchi per terra». Ebbene, da allora di buchi in Basilicata ne sono stati fatti 447, altro che quattro. L'abitudine di questo Governo a tenere sotto silenzio le questioni importanti e le grandi verità la riscontro anche nell'attività di alcuni dei suoi componenti, in particolare quelli lucani; e da lucano lo devo ribadire. Faccio riferimento, in maniera puntuale, al vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, che guarda caso qualche giorno fa, l'8 aprile, se n'è uscito con un'intervista nella quale parlava della questione di Tempa Rossa e dello scandalo

perché i protocolli di legalità, che dovevano garantire trasparenza, non sono stati rispettati. Ma di che sta parlando il Vice Ministro, come se fosse calato da Marte giusto l'altro ieri? Il vice ministro Filippo Bubbico è stato assessore alla sanità e all'ambiente dal 1995 e l'anno dopo, per altri cinque anni (quindi dal 2000 al 2005), è stato governatore della Basilicata; si tratta degli anni nei quali veniva firmato il protocollo di intesa tra ENI, Shell e Regione. Successivamente, nel 2006 in particolare, veniva firmato un *memorandum* tra Governo e Regione dal successivo governatore della Basilicata Vito De Filippo, guarda caso un altro componente di questo Governo, Sottosegretario alla salute. In quel protocollo si ribadivano i concetti che, se mi posso permettere di esprimerlo con una locuzione che uso abitualmente, caratterizzano questo Governo come un "Governo fossile". Infatti, signor Presidente, da quegli anni nella sede dell'ENI in Basilicata, che si trova nell'ex convento di Viggiano, si è assistito ad una processione continua di portatori di interessi, leciti e meno leciti, da far impallidire la processione che ogni hanno i fedeli fanno per portare la Madonna

E a proposito di pellegrinaggi - mi tocca dirlo in quest'Assemblea - quanto ancora devo aspettare, in termini di pellegrinaggi, perché la Commissione di inchiesta su ENI che ho chiesto a questo Senato a settembre 2015, anzi a giugno 2015, finalmente possa vedere la luce? Devo aspettare qualche pellegrinaggio in particolare? Di chi? Me lo dica, magari più tardi, il Presidente del Consiglio, che con il suo partito e con il Nuovo Centrodestra non fa che mettere i bastoni tra le ruote alla discussione e all'approvazione di questa Commissione di inchiesta su ENI, che noi vogliamo non perché intendiamo affossare l'azienda, ma perché ci vogliamo vedere chiaro su un patrimonio della nazione, che però è anche parte di uno scandalo che vede coinvolti cinque suoi dirigenti in Basilicata.

Ha 14 dighe, che hanno una capacità totale di più di un miliardo di metri cubi di acqua potabile. Ha sorgenti che erogano 10.000 litri circa al secondo, che sarebbero 600.000 litri di acqua buona al minuto, 864 milioni di litri al giorno e più di 315 miliardi di litri rinnovabili all'anno. Al contrario, questo Governo fossile, ma anche i precedenti, spinge per il petrolio presente nel sottosuolo lucano, che è valutato in circa 800 milioni di barili in totale. A confronto di 315 miliardi di litri rinnovabili di acqua buona gli 800 milioni di barili sono essenzialmente non rinnovabili, e non lo devo dire certo io, che sono un modesto geologo di provincia.

Per estrarlo, per perforare e per ricercarlo, si arriva ad utilizzare fino a 500 sostanze, molte delle quali tossiche e nocive, e alcune anche radioattive, come l'americio 241. di buchi, in Basilicata, dal 1997 a oggi, ne hanno fatti 447, e non i 4 di cui si diceva prima, e li hanno fatti a 500 metri da un ospedale, vicini alle aree di ricarica delle sorgenti, nelle case coloniche

a uno studio durato vent'anni, presentato dall'Istituto tumori di Milano, la Basilicata è risultata come una Regione che, dal 1990 al 2010, ha un tasso di incidenza tumorale con andamento doppio rispetto alla media nazionale. Quindi, in parole povere, in vent'anni la Basilicata ha raggiunto, nell'incremento tumorale, tutte le altre Regioni d'Italia. Cosa ha l'ex Presidente della Regione Basilicata, l'attuale sottosegretario alle salute Vito De Filippo? Per sminuire questo dato fece realizzare un'altra ricerca dall'Università La Sapienza, relativa solo all'anno 2010. Ovviamente, l'incremento era già avvenuto e nell'anno 2010 le percentuali tumorali in Basilicata risultarono di poco inferiori a quelle della media nazionale. Il governatore De Filippo ebbe allora la stessa uscita che ebbe Maria Antonietta d'Austria quando disse ai suoi sudditi pane, potevano mangiare le *brioche*. Egli diede la colpa allo sviluppo industriale, al fatto che anche le famiglie lucane avevano potuto mangiare un sacco di merendine e che era arrivato finalmente lo sviluppo anche in Basilicata. Questo è il comportamento politico delle persone che siedono in questo Governo: mistificare, sminuire, cancellare se va bene. E quindi, poiché si tratta di un sistema un sistema petrolio, che è oggettivamente un sistema di interessi economici, industriali, politici e molto spesso illeciti, dai quali il Governo non può ritenersi immune e neanche politicamente non responsabile per le connessioni che ha con detto sistema, chiedo all'Assemblea del Senato di votare la presente mozione ed esprimere quindi la sfiducia al sistema Governo nel suo complesso, cominciando dal suo astro, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, passando da tutti i pianeti che gli ruotano intorno, quali i ministri Boschi, Alfano, Padoan e gli altri, fino ad arrivare ai pianetini, quali il vice ministro Bubbico, e terminare con gli asteroidi, gli ultimi della fila, quale il sottosegretario alla salute

per diverse ragioni. La prima, quella che ci ha dato l'occasione, è la vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro Guidi, la quale ha ritenuto di doversi dimettere per la vicenda molto nota, finita sui giornali.

Non sarebbe così se fosse stato possibile un confronto punto per punto, in cui sul famoso emendamento di cui tanto si è parlato ognuno avesse avuto modo di esprimersi, anche nella maggioranza. Così non è stato e dunque la responsabilità è collettiva. Ricordiamo che quell'emendamento, poi passato nella legge di stabilità insieme ad altri 654 commi sui quali il Senato ha avuto modo di dire solo o sì a tutto o no a tutto,

adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza; se invece si vuole consultare qualcuno, forse bisognerebbe consultare il Parlamento, qualcuno altro e non solo i diretti interessati. Naturalmente non c'è solo questa vicenda specifica, c'è ben altro. Noi presentiamo questa mozione perché il PIL italiano registra un tasso di crescita tra i più bassi in Europa e presenta un effetto ottico per cui più è lontano e più cresce, mentre man mano che si avvicina la scadenza

al 3 per cento di PIL in meno rispetto al 2011, quando c'è stato l'ultimo Governo espressione diretta dei cittadini, l'ultimo votato e che si basava su maggioranze alle quali i cittadini avevano chiesto di sostenere questo Governo, a differenza del suo che è votato in modo significativo e decisivo da

80 euro di più in tasca, ma hai anche 80 euro di debito in più in banca. Tutti gli altri invece si sono semplicemente presi i debiti in più senza avere nessun beneficio, oltre a diverse tasse che sono aumentate.

signor Presidente del Consiglio, lei aveva promesso che entro il 21 settembre 2014 sarebbero stati pagati tutti i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Il 21 settembre è una data che le è molto cara, era diventata molto cara anche a tutte le imprese che aspettavano il pagamento. Purtroppo l'hanno pagata cara, perché il pagamento ancora oggi non è completato e tante imprese hanno chiuso, tanti posti di lavoro sono andati perduti perché non è stato rispettato questo preciso impegno. Ce n'è più che abbastanza, su ciascuno di questi punti, per votare la sfiducia, per chiedere a questo Governo di passare la mano perché già abbastanza danni ha fatto.

Io, visto come stanno andando ultimamente le cose in quest'Assemblea, sono invece un po' più realista, un po' più sfiduciato sulla mozione di sfiducia. di sfiducia. Oggi come oggi, venire in Aula, signor Presidente, e cercare di convincere i colleghi senatori della bontà della nostra mozione di sfiducia penso possa essere considerata una *mission impossible*.

Oggi come oggi, questo è solamente esercizio politico d'Assemblea per poter condividere e cercare di far arrivare, grazie agli organi di informazione, a più persone possibile, quanto sta facendo questo Governo. avrei potuto mettermi qui a parlare, a dire, a raccontare, a spiegare le motivazioni tecniche per cui questo Governo deve andare a casa.

del peggior comitato d'affari messo in un Governo della Repubblica italiana. Di conseguenza, siamo qui ad assistere ancora una volta a tutti i giochini e giochetti, Ministri che si dimettono, gente indignata, sostituzioni varie di persone che, se non ci fossero state le intercettazioni telefoniche, le avremmo viste ancora sorridenti nei banchi del Governo. In una legislatura - sono qui da pochi anni - in cui è vero che il Presidente del Consiglio è cambiato, ma la maggioranza, alla fine, è più o meno la stessa, noi ci siamo trovati tante persone che siedono in quei banchi che hanno avuto pruriti da parte della giustizia: penso al ministro Cancellieri, all'ex ministro Idem, all'ex ministro Lupi, a tutte le famiglie Boschi, Renzi, Lotti, a tutto quello che è successo, di cui abbiamo già parlato in queste Aule e su cui abbiamo letto chilometri e chilometri di parole sui giornali; anche all'ex ministro Guidi, all'ex membro del Governo De Filippo. Quindi ne abbiamo visti e temo che ne vedremo, perché, come ben sappiamo, questa mozione di sfiducia

Nelle scorse ore ero a Latina. Per la campagna elettorale ci siamo fatti due giorni a Latina e abbiamo incontrato centinaia di cittadini e con tutti abbiamo parlato di cose serie e importanti. Abbiamo parlato di riforma Fornero, quella maledetta riforma che buona parte degli italiani vorrebbero rimandare al mittente. Abbiamo parlato di immigrazione, sicurezza e lavoro, tutte problematiche che con questo Governo non si riescono a trattare

da persone che sono state elette con i voti degli elettori del centrodestra, persone che, in buona fede, sulla scheda elettorale avevano messo una croce

avremo ancora questo Presidente del Consiglio e questo Governo. Prepariamoci perché ottobre non è così lontano: una bella estate di vacanza e poi lo mandiamo a casa.

Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, non parlerò in questi cinque minuti del merito dell'inchiesta di Potenza. Innanzitutto perché non la conosco abbastanza, poi perché i giudizi penali non si danno in questa Assemblea e, infine, perché le garanzie valgono per i propri avversari ancora prima che per gli amici. Io questa regola l'ho sempre rispettata e non verrò meno oggi, anche perché questo mi consente di evidenziare il modo distorto con il quale il Presidente del Consiglio fa professione di garantismo. del Consiglio, questa vicenda ha reso ancora più oscura di prima, se è possibile, la categoria dell'opportunità politica che ha fin qui guidato il suo approccio Grazie a tutte l'ennesimo, dimettersi per opportunità politica a seguito di un'intercettazione riguardante un emendamento del Governo; il giorno dopo il *Premier* assumersi la responsabilità di quel testo: "l'emendamento *c'est moi!"*; in seguito si è appreso del coinvolgimento nell'inchiesta di un Sottosegretario, stavolta come indagato e in nome della presunzione d'innocenza il problema non è stato proprio posto. Io sono sempre stato contrario - e rimango contrarissimo - all'automatismo per cui l'iscrizione sul registro degli indagati debba comportare obbligatoriamente le dimissioni. Ciò, infatti, significherebbe demandare agli inquirenti la selezione della classe politica prima ancora della celebrazione di un processo e privare così la politica della sua autonomia. Ma mi sembra che ormai siamo al paradosso per il quale, per evitare le dimissioni, si debba attendere l'avviso di garanzia. Se non sono indagato la mia sorte è appesa alla categoria dell'opportunità politica, applicata con una certa - diciamo

La seconda antinomia che questa vicenda evidenzia riguarda la legislazione e le sue conseguenze. Proprio in nome di quella separazione dei poteri tanto evocata, che assegna ai legislatori il compito di scrivere le leggi e ai magistrati quello di applicarle, non si può adottare una legislazione che giurisdizionalizza tutto e segmenta le fattispecie rincorrendo i fenomeni sociali - pensiamo ai reati ambientali, al femminicidio, all'omicidio stradale - e poi e poi lamentarsi perché i magistrati si adeguano all'approccio dei legislatori. Non si può introdurre nell'ordinamento un reato evanescente come il traffico di influenza in assenza di una regolamentazione dell'attività di *lobbying* tanti colleghi in quest'Assemblea, quelli presenti anche nella scorsa legislatura, ricorderanno quanta fatica ci costò fissare quantomeno il parametro del vantaggio patrimoniale indebito - e poi lamentarsi se l'attività inquirente finisce per lambire la sfera della decisione politica. Infine, signor Presidente del Consiglio, da un Capo di Governo ci si aspetterebbe almeno un po' di precisione. Infatti, con l'abilità retorica che certo non le manca, credo che per difendere il Governo su Tempa Rossa lei abbia creato una intenzionale confusione comunicativa tra opere pubbliche e iniziative private. Sia chiaro che contro queste ultime

che la Total non è l'ENI. Un ripasso delle vicende libiche degli ultimi anni forse aiuterebbe a mettere un po' meglio a fuoco la differenza. Non si può infine accusare i magistrati di non giungere mai a sentenza e poi - al di là della sfortuna di averlo fatto poche ore prima di una sentenza invece di pensare a come deflazionare il sistema penale, da una parte si allunga ancora la prescrizione del reato senza prevedere la prescrizione del processo, e dall'altra si devolve ai giudici perfino l'autocertificazione per il canone RAI. Signor Presidente, per tutte queste ragioni noi non avremmo presentato una mozione di sfiducia, ma, per tutte queste ragioni, di fronte a una mozione di sfiducia, voteremo a favore. Signor Presidente, colleghi, queste mozioni di sfiducia sono la conferma, purtroppo, di una concezione della politica come delegittimazione dell'avversario politico di turno. Pensavo che, dopo vent'anni di berlusconismo e di antiberlusconismo che hanno stremato il nostro Paese, potesse sorgere una fase politica nuova, in cui poter mettere dietro le nostre spalle la permanente contrapposizione e inaugurare un nuovo modo di concepire il confronto politico, fondato sul merito e sul rispetto reciproco. Invece, dal comitato di liberazione contro Berlusconi siamo passati al comitato di liberazione contro Renzi, formato da tutte le opposizioni, compresa quella parte politica di cui ho fatto parte anch'io, che ha subìto per vent'anni un'opera incessante di delegittimazione politica e morale. Siamo immersi nello stesso clima e nella stessa atmosfera di odio che una certa disinformazione mediatica alimenta quotidianamente, e del connubio fra indagini giudiziarie e divulgazione di intercettazioni telefoniche, che formano una miscela di sfiducia verso tutti e verso tutto. La Sinistra dei girotondi è stata sostituita dal Movimento di Grillo, il cui antagonismo preconcetto verso qualunque decisione del Governo è condiviso oggi dalla nuova Lega lepenista in nome di un nazionalismo che confligge sia con il federalismo che con l'europeismo. Ci chiediamo che cosa sia successo al centrodestra; è come se fosse andato a lezione di giustizialismo da Marco Travaglio, a lezione di costituzionalismo dai *fan* della "Costituzione più bella del mondo", a lezione di decrescita felice dai teorici dell'anti-industrialismo. In ogni caso, è per tutte queste ragioni che oggi tutto l'arco delle opposizioni si ritrova a sostenere nuove - le ennesime - mozioni di sfiducia nei confronti del Governo, sulla base di pretesti che potrebbero essere invocati ogni giorno per sfiduciare un Governo in carica. L'obiettivo, tuttavia, non è quello di sfiduciare il Governo, che gode di un'ampia maggioranza, né quello di indicare un progetto alternativo di governo, che con tutta evidenza non esiste. L'obiettivo vero, comune a tutte le forze di opposizione, è quello di negare l'evidenza, e cioè che finalmente c'è un cambiamento in atto; l'obiettivo vero è quello di tentare di annullare, con una polemica spinta al massimo della falsificazione, ogni risultato positivo concreto ottenuto da questo Governo. Si spiegano in questo modo persino, purtroppo, gli attacchi irrispettosi - fino al vilipendio - nei confronti del Capo dello Stato, a cui va tutta la nostra convinta solidarietà, e perfino nei confronti del Papa, trattato alla stregua di un qualunque politico. Insomma, coloro che oggi voteranno insieme la sfiducia al Governo sono uniti solo dalla volontà di creare il massimo della confusione, il massimo della sfiducia, il massimo della rabbia contro chiunque abbia responsabilità di governo, a livello nazionale e internazionale, e operi secondo un'idea democratica per governare il mondo, squassato oggi da tante tensioni e sfide inedite. Le mozioni di sfiducia verranno respinte, cari colleghi - lo sappiamo tutti - ma coloro che le sostengono continueranno nel loro gioco al tanto peggio tanto meglio, continueranno a soffiare cinicamente su tutte le tragedie del nostro tempo, continueranno ad alimentare tutte le paure e le preoccupazioni, in parte comprensibili, ma con l'unico scopo di lucrare consensi sulle sofferenze e sulla pelle della gente, e sui problemi epocali che sono di fronte a noi e che richiederebbero invece un confronto serio, con soluzioni serie e praticabili. Ben vengano perciò queste mozioni di sfiducia se servono a mostrare qual è la posta in gioco, qual è la differenza fra le due Italie che esistono c'è l'Italia che, consapevole delle molte difficoltà accumulate nel tempo, agisce concretamente per risolverle; e purtroppo c'è un'altra Italia, che punta sulle divisioni,

quella che, nonostante tutto, vuole essere positiva, vuole guardare al futuro, ad un mondo che ha anche bisogno di noi - come ha detto il nostro *premier* Renzi - ad un mondo difficile e complicato, ma che al tempo stesso può offrire tante opportunità, soprattutto ai giovani. Anche per questo diciamo no alle vostre mozioni di sfiducia, perché voi non rappresentate alcuna alternativa seria; non rappresentate nessun futuro migliore. Siete solo l'espressione dell'irresponsabilità, dell'incapacità di cambiare e del fallimento.

rappresentanti del Governo, ho una manciata di secondi per esprimere alcune brevi considerazioni su quanto siamo chiamati a discutere e votare quest'oggi. Mi preme sottolineare che Italia dei Valori ha apprezzato le dimissioni del ministro Guidi, un atto dovuto a seguito di una vicenda deprecabile, mentre non si può dire che sia apprezzata allo stesso modo la politica energetica di questo Governo. Ancor di più, abbiamo provato stupore, incredulità e anche irritazione di fronte agli inviti all'astensione dal voto referendario o alle legittimazioni del non voto, provenienti da persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi istituzionali di primo piano. Sia chiaro: l'astensione è un comportamento costituzionalmente corretto, votare ai *referendum* è frutto di una scelta libera. Prevedendo un *quorum* di partecipazione, l'articolo 75 della Costituzione riconosce la non partecipazione al voto come una volontà legittimamente espressa. Il voto però è un dovere morale. Italia dei Valori si è schierata per il sì al *referendum* e per il sì al rispetto dello strumento costituzionale referendario, che si manifesta in primo luogo partecipando al voto. Non possiamo quindi certo essere accusati di avere una posizione accondiscendente o missionaria nei confronti di un Governo che contrastiamo, invece, ogni qual volta le sue scelte si allontanano dai nostri valori e dalle nostre idee. Se dovessimo quindi votare solo e soltanto sull'oggetto principale delle mozioni oggi in discussione, laddove si chiede di esprimere un giudizio sulla vicenda del ministro Guidi e sulle ombre di conflitti d'interesse diffusi che aleggiano sul Governo, come Italia dei Valori, coerentemente con le nostre battaglie e i nostri principi, ci esprimeremmo a favore delle mozioni di sfiducia. Se dovessimo dare voce solo alla pancia, o forse anche al cuore, senza pensare alle conseguenze e senza pensare al bene dell'Italia, voteremmo a favore. Ma la mozione di sfiducia esprime un giudizio complessivo, è un atto politico foriero di conseguenze che non possono essere ignorate da chi vuole svolgere la propria funzione nell'interesse della Nazione. E allora dobbiamo constatare, ancora una volta, che non esiste in questa legislatura un'alternativa di Governo possibile, più vicina ai nostri valori e alle nostre idee rispetto al pur non sempre soddisfacente Governo Renzi. Esistono progetti di legge essenziali che devono essere portati a termine. Esiste una situazione economica e politica internazionale che necessita di stabilità di Governo. Le alternative, se c'erano, andavano trovate prima. Adesso, nel bene e nel male, dobbiamo quantomeno arrivare ad ottobre. La crisi politica Europea, Shengen, il rischio Brexit e l'eterna questione Grecia sono tutte bombe ad orologeria con le quali non possiamo scherzare per speculazioni politiche. E poi ci sono questioni sul tavolo ancora aperte, cui, come Italia dei Valori, crediamo e siamo fortemente interessati e nei confronti delle quali il Governo Renzi ha dimostrato di essere un interlocutore valido: la legge sulle unioni civili, l'ottava salvaguardia per gli esodati, la fattibilità di interventi volti a favorire una maggiore flessibilità nelle scelte individuali, per andare in pensione, la revisione dei lavori usuranti, il riconoscimento alle donne dei carichi di lavoro familiari, sono solo esempi di buon lavoro e buoni progetti da portare a termine. Per non parlare del caos che deriverebbe, in questo momento, dall'ipotesi di elezioni anticipate: con una legge elettorale alla Camera su cui pende già la spada di Damocle del giudizio della Corte costituzionale, una legge per il Senato neppure votata ma frutto di una sentenza, e delle riforme costituzionali in attesa di voto referendario. Non è possibile, quindi, esprimere un giudizio su questa discussione senza tenere conto, responsabilmente, dell'attuale assenza di alternative migliori al Governo di Renzi e del Partito Democratico. Nonostante non sia una grande statista

Signor Presidente, parto da una premessa: le due mozioni di sfiducia sono entrambe ispirate, suggerite e argomentate sulla base di illecite indiscrezioni di atti segretati, non essendo concluse le indagini in corso. Va osservato che questa premessa non è ininfluente su quello che stiamo facendo tutto quello che è stato divulgato e propalato, dobbiamo dirlo, o non riguardava persone indagate, sottoposte ad indagini, o comunque non doveva essere reso noto proprio perché le indagini erano in corso. Sulla base di questa premessa vorrei brevemente sviluppare i miei modesti concetti. Credo che tutti noi riconosciamo l'attività legislativa pienamente lecita in una democrazia rappresentativa, il processo di legiferazione, l'ascolto degli interessi organizzati, il dialogo con i cittadini, sia come singoli, sia come associazioni, sia come imprese, non solo è ammesso, ma è necessario e doveroso. Vorrei richiamare la mia personale esperienza nel Parlamento europeo, dove sono stato per nove anni. Nel corso del mio primo mandato ero vice Presidente della Commissione trasporti e sono stato il primo relatore - nel senso che

le associazioni dei disabili, quelle dei trasportatori, gli interessi organizzati di parecchi Paesi, sia di singole imprese che di organi di dimensioni più aggregate. Addirittura sono arrivati a suggerirmi esplicitamente alcuni emendamenti, che in parte sono stati accolti e in parte rifiutati a seconda dell'apprezzamento che poteva essere dato per arrivare ad un'unità ragionevole di un provvedimento così importante che avrebbe riguardato il modo di viaggiare di 550 milioni di europei. europei. Ora, stiamo parlando di una mozione di sfiducia che si basa su argomenti di per sé leciti che sono stati stravolti da una comunicazione fuorviante e da indagini che non si sa fino a che punto arriveranno ad una conclusione di condanna e che quindi, con la riserva che la Costituzione ci consente, sono da considerarsi perfettamente leciti.

guardasigilli. Il magistrato che aveva sviluppato queste indagini, poi conclusesi con il nulla, è diventato sindaco di Napoli e prima deputato europeo

noi oggi voteremo contro la sfiducia e a favore, quindi, del Governo in carica, ma questo aspetto, la fiducia al Governo, diventa secondario rispetto al fatto che noi oggi non votiamo tanto o soltanto la fiducia al Governo, votiamo la fiducia del Senato della Repubblica - ancora della Repubblica e non delle autonomie locali - verso i principi della Costituzione repubblicana che prevedono la separazione dei poteri. E se la magistratura, com'è giusto che sia, è indipendente nell'assumere le proprie decisioni, nel fare le proprie indagini e nell'emanare le proprie sentenze, il Parlamento della Nazione è libero e indipendente di legiferare, di compiere gli atti legislativi necessari al Governo e il Governo ha il dovere di scegliere e di adottare le decisioni più appropriate.

Solo la Costituzione può dirci che le leggi che facciamo sono improprie, non una procura, né un tribunale ordinario e lei lo sa bene, Presidente, perché viene da quella Mi avvio rapidamente alla conclusione: sulla base di questi motivi che non sono solo del Governo, ma sono della Repubblica italiana, noi confermiamo una fiducia che non può essere tolta per atti che partono da illecite propalazioni di documenti e che non hanno alcun riferimento alla sostanza della nostra istituzione repubblicana. *(CoR)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, le mozioni di sfiducia rientrano nelle normali dinamiche parlamentari e contrappongono maggioranza e opposizione. Nella presente legislatura, la maggioranza che guida il Paese ha votato cose ben più scabrose e sono perciò convinto che, anche questa volta, il Governo Renzi avrà strada libera. Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti, senza molto coinvolgimento, voterà comunque la sfiducia. Dico così perché questo voto rimarrà un episodio fine a se stesso, una pura esercitazione di posizionamenti politici

il dramma della salute pubblica, insomma, ed è un dramma vero, che si respira, che la nostra popolazione comincia a comprendere e che io, come parlamentare della Basilicata, ho il dovere di denunciare in questa una piccola Regione, ma ha il più grande giacimento di petrolio *off-shore* dell'Europa occidentale. Ogni giorno, nelle viscere di quella Regione, viaggiano 3,4 milioni di metri cubi di gas e 81.868 barili di petrolio: per inciso, un barile contiene 159 litri di petrolio. Che ne dite? Non è male come patrimonio. Un

studi e ricerche, che in materia di trivellazioni significano salvaguardia ambientale e che pongono quel Paese all'avanguardia a livello mondiale, un fondo sovrano gestito dalla banca centrale, ma di proprietà del Ministero delle finanze, diventato il fondo più grande del mondo, che possiede l'1 per cento del mercato azionario mondiale e innumerevoli proprietà in giro per il mondo.

cento, in cui ci sono uno dei migliori *welfare* al mondo, sussidi per i giovani meno fortunati, 40 miliardi di avanzo primario annuo e il terzo PIL più alto al mondo. nella "Basilicata Saudita", come la chiama il mio amico Maurizio Bolognetti, segretario dei radicali lucani e memoria storica dei disastri ambientali provocati dalle perforazioni? I numeri della "Basilicata Saudita" sono a dir poco imbarazzanti per una classe dirigente che tale si voglia chiamare. Il reddito *pro capite* è il più basso d'Italia, la disoccupazione giovanile è intorno al 50 per cento, le infrastrutture sono inesistenti signor Presidente del Consiglio, basta citare Matera, capitale europea della cultura, unico capoluogo di provincia italiano non ancora raggiunto dalle Ferrovie dello Stato *(Commenti del senatore Può bastare? Basterebbe anche. È che purtroppo sembra di rileggere il resoconto di Manlio Rossi Doria, economista e grande meridionalista, quando scriveva, confinato in Val d'Agri dal fascismo, che la miseria contadina dal petrolio non trae alcun beneficio. Non siamo più a quei tempi, né alle citazione folcloristiche di Marcello Sorgi. A proposito: non ho ancora compreso se sparare così tante imbecillità aiuti a diventare direttore del TG1 o serva a farsi ospitare nei salotti televisivi. Ma torniamo alla Basilicata, terra meravigliosa e ricca di storia, di cultura, di tradizioni e di risorse naturali: acqua, petrolio e gas innanzitutto. 550.000 abitanti dovrebbero essere ricchissimi e invece sono i più poveri, ma quel che è peggio è che sulla meravigliosa terra della Basilicata, conosciuta anche ai tempi dei romani come il granaio d'Italia, incombe la minaccia di un disastro ambientale. Questo perché, come scrive il procuratore nazionale antimafia, il distorto connubio tra imprenditoria e politica ha prodotto una organizzazione criminale che lucra su tutte le imprese e le lavorazioni del petrolio. E come? Dividendosi appalti, taroccando codici, occultando analisi e monitoraggi ambientali, avendo cioè, come strada maestra, l'intrallazzo e la menzogna. Volete qualche prova? Gli ultimi tre presidenti di Confindustria Basilicata lavoravano e lavorano avendo come principale cliente la Regione Basilicata. Uno addirittura, per non farsi mancare nulla, ha anche accettato di fare l'assessore regionale alla sanità. La sanità, appunto. Sapete a cosa servono le *royalty* del petrolio? A pagare la sanità pubblica, quella regionale, dove, se non hai la tessera del Partito Democratico, non puoi fare nulla, né l'infermiere, né il medico, né il direttore sanitario.

un intreccio perverso, questo sì fermo ai tempi di Banfield, quando, dopo nove mesi di studio a Chiaromonte, un paesino della Lucania, nel 1958 pubblicò il libro «The moral basis of a backword society», cioè la storia del familismo amorale. La Basilicata purtroppo questa perversa politica ce l'ha ancora tutt'oggi; è una perversa politica che regola e dirige tutto, tutto impregnando di sé. Tutti famigli, dalle ASI alle APT, passando per l'ARPAB, l'ARBEA e i Consorzi di bonifica; insomma, tutto quello che è regionale. Un reticolo dove controllati e controllori appartengono alla stessa famiglia, alla stessa scuola, alla stessa cultura; la cultura di quelli che sfruttano i bisogni della gente. Ed è così che la grande ricchezza di pochi ha generato la povertà di molti. Tutto questo sotto la regola aurea della menzogna. Ti rubano la vita e la libertà e, in cambio, ti promettono un posto di lavoro che difficilmente arriverà. E distribuiscono a pioggia i fondi delle *royalty*, sponsorizzano sagre, fiere di paese, feste patronali, incontri di circoli e bocciofile. La beffa, dunque: ridi, ti diverti, non pensi a nulla e diventi povero. E, se sei sfortunato, ti ammali pure. Servo sei e servo devi rimanere: la regola aurea del partito dei lavoratori. Ben vengano allora uno, mille, centomila fidanzati di Ministri, se le loro storie servono ad alzare il velo su uno dei più terribili scandali della politica italiana. Uno scandalo vero, non immaginato da gufi o da quelli che remano contro lo sviluppo del Paese, del quale, speriamo presto, la magistratura ci definirà i contorni veri. Presidente, onorevoli senatori, poco fa ascoltavo qualche commento giornalistico all'esterno dell'Aula

materiali e concrete, ancorché politiche, che hanno portato a presentarle. Ormai ci siamo abituati un po' a queste cortine fumogene, per cui alla fine si sposta l'attenzione dell'opinione pubblica e quasi si fa passare questa come un'iniziativa che fa perdere al Governo il suo abbrivio di operosità, che vorremmo però fosse in direzione quantomeno onesta e in direzione quantomeno certa degli interessi dei cittadini. perché ricordiamo che, se siamo arrivati a queste mozioni di sfiducia, non è perché le opposizioni sono brutte e cattive, ma perché c'è un Governo composto da gente che è stata chiamata a ricoprire incarichi di Ministro e che si è macchiata di atteggiamenti al limite dell'offensivo nei confronti dei cittadini. Gente che perde o che non ha il posto di lavoro e poi legge dai giornali di intrallazzi fatti per collocare l'amico di partito da una parte o dall'altra. Cittadini che fanno fatica ad arrivare a fine mese e poi leggono dai giornali di discorsi tra il Ministro e il suo compagno che a tutto attengono fuorché alla sfera dell'interesse pubblico. Diciamolo perché siamo arrivati a questa mozione: perché non possiamo essere governati da un Governo composto da gente corrotta! Questa è la verità dei fatti!

e interessi di Governo, che dovrebbero essere invece indirizzati al Paese. Vede, presidente Grasso, il Governo sta soffocando in maniera vistosa nei rapporti lobbistici con cui si sta finanziando la politica di chi sostiene il Governo. E sono questi rapporti lobbistici che stanno mandando al macero il nostro Paese. Mentre il presidente Renzi, quando ha preso le redini del Governo, ha voluto dichiarare in discontinuità rispetto a un passato di politiche inconcludenti, che al nuovo Esecutivo interessava che la politica fosse fatta da gente che lavora nell'interesse dei cittadini. E invece quanto è emerso nei rapporti tra il ministro Guidi, i suoi collaboratori e le *lobby* non è nell'interesse dei cittadini. Su questi punti bisogna essere chiari. Cosa accadrà oggi? Verrà votata la mozione di sfiducia. Il Governo avrà la fiducia o non avrà la fiducia? Lo vedremo tra poche ore. Una cosa è sicura: avremo la certificazione, per l'ennesima volta, di chi compone la maggioranza su cui si regge il Governo. Perché piaccia o non piaccia a quella minoranza del PD, che tanto poi si fa spavalda quando si mette alla tastiera, quando va su Facebook o su Twitter, il Governo Renzi non lo reggete voi, ma lo reggono AL-A, Verdini e la sua maggioranza!

Non dovreste piegarvi a questi interessi e dovreste oggi votare la sfiducia al Governo. Fate pulizia! Lo dico anche a qualcuno che magari ha paura. Non abbiate paura di tornare al voto, perché nel voto c'è solamente un momento di democrazia

Se infatti il Paese reagisce in maniera rabbiosa, è quella che i cittadini si stanno facendo di questo Governo è un'opinione che attiene ad aggettivi come trafficoni, maneggioni, intrallazzoni, sfacciati, imbroglioni e disonesti. E un Governo che non è onesto non può governare il Paese e non può essere di esempio agli altri cittadini che in maniera onesta e corretta pagano le tasse. Questa è la ragione per la quali oggi ci si trova qui a votare la mozione di sfiducia. Perché siete degli intrallazzoni, e noi non vogliamo un Governo di intrallazzoni! Vergognatevi!

Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve e anche molto più pacato, perché le due osservazioni che intendo proporre all'attenzione del Governo

che finisce nel mirino di una mozione di sfiducia per una questione di trasparenza. Questo è oggettivo. È la prima volta che in Italia un Governo, di sinistra o di centrosinistra, che dir si voglia, si voglia, viene chiamato in causa in un dibattito parlamentare per una questione di trasparenza. Questo è un fatto statistico importante - e lo vorrei sottolineare anche nei confronti

che anche a sinistra è serio il problema di far progetti di potere, che anche a sinistra c'è una dinamica per cui il confine tra l'interesse pubblico e quello di *lobby* e di parte

naturale: le persone sono fatte di attese, tensioni, pulsioni che le rendono identiche. In questo senso mi permetto di rovesciare il ragionamento che faceva la collega Repetti. Certo, giustamente per venti anni si è detto c'era una tendenza a criminalizzare i Governi di centrodestra, quasi che centrodestra significasse di per sé malaffare. Tuttavia questo ragionamento è cominciato ben prima,

cioè ad un'interpretazione della storia dove il racconto dei vincitori, o di quelli che in quel momento sono preponderanti, inchioda chi invece vuol fare politica con un progetto magari parziale, ma comunque che mira al bene per il Paese. La seconda caratterizzazione della mia riflessione è politica.

né forse una *leadership* realmente propositiva per essere realmente competitiva. Da questo punto di vista, quindi, lei è tranquillo. Ha solo un problemino, un ospite indesiderato a cena che si chiama realtà,

questa repulsione che il Governo ha nei confronti della realtà, ci convince che ogni occasione è buona, non per dare una spallata, ma perché la gente si accorga di ciò che è vero. E cosa è vero? Pochi giorni fa il Governo ha siglato un accordo tra l'Unione europea e la Turchia sul tema della migrazione. Forse non ha letto le carte, perché siglare un accordo in cui il Mediterraneo

all'Italia di non essere vittima predestinata di quello che accade nell'area Sud del Mediterraneo è un sintomo chiaro di come la realtà non sia quella che viene raccontata. Infatti, in realtà l'Italia, laddove deve contare, non conta;

che mette in evidenza la presenza di una tensione positiva, perché nel procedere del tempo, goccia dopo goccia (ma è una goccia che scava la pietra) inevitabilmente il destino italiano appare compromesso. al provvedimento sulla buona scuola. Vi siete accorti del caos che c'è nelle scuole italiane? Vi siete accorti di aver trasformato il cosiddetto organico aggiuntivo degli insegnanti in una masnada di persone che non riesce ad essere impiegata con senso compiuto? Vi siete accorti che molte delle misure che avete varato non sono repulsive perché erano sbagliati i titoli, ma più semplicemente perché avete scritto malissimo i capitoli? È per questo che esprimo tutta la mia comprensione verso le persone coinvolte in queste sciagurate vicende paragiudiziarie, soprattutto in particolare verso il qui presente sottosegretario De Vincenti. Io auspico che un giorno possano essere pubblicate le mie intercettazioni. Sono certo di aver avuto sempre, nei suoi confronti, signor Sottosegretario, ma anche di qualunque rappresentante del Governo, espressioni molto più lusinghiere ed affettuose.

dell'Italia e che intende seguire chiunque abbia un progetto di riforme liberali. Prima lo abbiamo fatto con il presidente Berlusconi, e adesso lo stiamo facendo, credo da pretoriani, con il suo Governo, signor Presidente. Invero, la nostra storia, la mia e quella di altri colleghi, viene dalla Prima Repubblica: io sono socialista e prima o poi dovremmo dirci, nella parabola di Luca, chi è il figliol prodigo, chi è che è uscito e chi è che è entrato, ma questa sarà una discussione più politica che faremo. Siamo un Gruppo che ama ed esalta la mentre altri non l'apprezzano, la dimenticano, forse nemmeno la conoscono. Confesso di non sopportare l'atteggiamento di Gruppi politici che si vantano di non conoscere quello che è successo quando non erano ancora nati. Anch'io non ero nato ai tempi di Turati, ma lo conosco benissimo. Siamo un Gruppo, signor Presidente, che considera l'esperienza una virtù, mentre gli altri la considerano un danno, anche se poi ci si accorge che i dilettanti allo sbaraglio, quelli che la politica non la conoscono, che provengono dalla società civile, possono provocare anche danni al Governo, perché generalmente hanno anche un po' troppi parenti e fidanzati. Concludo, signor Presidente, dicendo che ben dicendo che ben si presta una canzone degli Squallor, ben interpretata da Rosanna Fratello, intitolata «Sono una donna, non sono una santa». La debolezza umana è anche questo; il male è che gli avvoltoi strumentalizzino questa debolezza umana. Ma in politica e nell'amministrazione oltre all'onestà ci vuole preparazione, capacità e coraggio. E noi, signor Presidente, riconosciamo queste doti nel suo Governo, ed è per questo che tutto il Gruppo unanimemente voterà contro la mozione di sfiducia.

sono da sempre garantista e da sempre convinto che i processi si fanno in tribunale, su questioni specifiche, per responsabilità soggettive e circostanziate, e non in Parlamento come si vuol fare oggi, né sui *media* (TV, giornali e Rete), come si fa di solito. Questi atteggiamenti sono praticati nei regimi peronisti, populisti, illiberali, autoritari. Signor presidente Renzi, devo ammettere che l'uso delle mozioni di sfiducia ripetute e strumentalizzanti, verso il suo Governo

per il perdurare di atteggiamenti improntati al pregiudizio e ad un'azione di opposizione strumentale, senza concrete proposte da buona parte di chi si oppone, il cui atteggiamento è spesso confondibile con comportamenti da saltimbanchi e da circo, che sfuggono costantemente al dovere della proposta e ad una contrapposizione sul merito, essendo solo capaci di critiche

a dare all'Italia efficienza, rapidità di decisione, riduzione dei burocratismi inutili e assunzione di responsabilità piena di quanti sono chiamati ad operare e a decidere. mi sono dovuto ricredere e mi sono dovuto convincere che il suo è un metodo efficace nella condizione data, giusto. I risultati sin qui raggiunti sono importanti, seppur non esaustivi, ma vale la pena elencarne alcuni: il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, varato con la riforma del ministro Madia, che sta affrontando decennali problemi di immobilismo è sinceramente un buon punto di partenza. Bisogna insistere, abbinandolo a una verifica impietosa e senza reticenze dei risultati positivi, ma anche delle distorsioni, con valenze perverse e penalmente rilevanti, prodotte dalla legge Bassanini sugli enti locali. Importanti passi in avanti sono stati fatti per il superamento di inaccettabili ritardi, privilegi, contraddizioni palesi, inadempimenti costituzionali nel settore della giustizia. Si sono raggiunti con gli interventi legislativi nei settori penale e civile che hanno concorso al miglioramento dei rapporti tra cittadino e sistema giudiziario. Voglio ricordare, come simbolo di un cambiamento di rotta, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che da decenni aspettava di essere resa effettiva con le modifiche introdotte. Presidente Renzi, oggi, però, dobbiamo colmare l'inaccettabile ritardo che abbiamo su unioni civili e testamento biologico, ed è necessario un diritto di famiglia più avanzato e - mi permetta, avendo in mente l'inaccettabile vicenda del nostro concittadino Giulio portare a termine la legge che introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano. Grandi passi in avanti sono stati fatti nella scuola pubblica con stabilizzazione degli insegnanti e responsabilizzazione dei dirigenti. Bene, così come bene si sta facendo nel campo della valorizzazione e promozione delle nostre ricchezze artistiche, culturali, ambientali e storiche che danno linfa al turismo e all'economia del nostro Paese. Vedo segnali più tenui nelle politiche economiche, ma sono consapevole delle difficoltà e dei pesi che derivano dal passato e dai vincoli internazionali presenti, ma so che il suo impegno e quello del suo Governo in questi campi sono forti. ultime considerazioni. La prima è sulla nostra politica europea ed estera: prudenza, ma anche determinazione, e vedo che lei si muove con questa impronta. necessario uscire dalla subordinazione, proporre, saper ascoltare e confrontarsi. È essenziale uno stimolo forte nei confronti della famiglia socialista europea, presidente Renzi, che purtroppo è troppo subordinata alle esigenze di politica interna. I socialisti hanno sempre saputo guardare lontano nel tempo e nel mondo; oggi lo stanno facendo troppo poco e lei fa bene a fare il battistrada nel richiamare tutti a un diverso impegno per affrontare il fenomeno epocale, e con tratti tragici, dell'immigrazione, per la pace nel mondo e, in particolare, nel Mediterraneo e in Libia, dove il nostro impegno deve essere significativo, determinato, ma scevro da semplificazioni e interventi muscolari. L'ultima questione riguarda le riforme costituzionali, di cui l'Italia ha un urgente bisogno. Mi consenta di dirle che si dovrebbe ampliarne l'ambito: non possiamo limitarle a quanto già fatto, e cito qualche titolo: riordino dei confini regionali ed eventuali accorpamenti; superamenti della frammentazione delle amministrazioni territoriali, Comuni in primo luogo; riforma del Consiglio superiore della magistratura, superamento dell'obbligatorietà dell'azione penale (che è rimasta una norma inapplicata) e separazione definitiva ed effettiva delle carriere. A proposito di separazione, incompatibilità e conflitti di interesse, ho perso di vista le proposte di legge che regolamentano queste materie particolarmente critiche nel definire gli equilibri tra i poteri, con particolare riferimento alla eleggibilità e incompatibilità dei magistrati. In conclusione, signor Presidente del Consiglio, si proceda con coraggio e visione lunga e, da questo punto di vista, mi permetta di fare un'aggiunta a quanto sin qui richiamato, oltre all'apprezzamento per l'azione intrapresa finalizzata a portare a conclusione rapidamente le grandi opere pubbliche incompiute che da anni sono la testimonianza della irresponsabilità di tutti, governanti e oppositori. Le suggerisco il varo di un significativo piano casa, non necessariamente di nuove costruzioni, per dare risposta alle centinaia di migliaia di famiglie che vivono nel disagio per l'assenza di una decorosa abitazione e di prendere una decisione definitiva e non altalenante sul Ponte di Messina, che deve essere realizzato, e senza il quale il Sud, la Calabria e la Sicilia rimangono territori separati, di fatto, dallo sviluppo che, seppur lentamente, sta ripartendo nel resto Presidente Renzi, avanti, guardi avanti e lontano. Noi siamo al suo fianco. Lei e il suo Governo avete la nostra fiducia.

poi, ha un'idea della democrazia che è, a dir poco, ottocentesca. La controriforma del lavoro e la controriforma costituzionale sono l'emblema di quanto affermo e io, da lucano e da operaio metalmeccanico, mi posso permettere di dirglielo. Lei ha distrutto il mondo del lavoro, ha distrutto il lavoro come bene sociale, come bene primario. Presidente Renzi, a proposito di democrazia, lei sta governando con la metà dei voti che il *referendum* antitrivelle ha raggiunto (16 milioni di voti, 14 milioni di sì): i voti che il Partito Democratico ha preso alle elezioni politiche del 2013 sono 8,6 milioni e per giunta con un programma elettorale che si chiamava «Italia. Bene comune», che lei ha trasformato in «Italia bene per pochi intimi e potenti». Lei deve spiegare politicamente, e non con chiacchiere da bar sport, dove - lo riconosco - lei è un fenomeno, come mai in Basilicata si estrae l'80 per cento del petrolio nazionale

Le ricordo che in Basilicata si estraggono mediamente 85.000 barili di petrolio al giorno, per non parlare del gas. L'unica cosa che ci avete portato è stato l'aumento delle malattie tumorali. Presidente Renzi, noi in Basilicata abbiamo tante eccellenze, al di là di quello a cui in questi giorni abbiamo assistito in TV e anche delle sue affermazioni. E la invito a riflettere quando parla di «quattro comitatini» e compagnia bella. La Basilicata ha delle eccellenze e, se vuole, gliele elenco tutte, a partire dall'Aglianico del Vulture, un vino eccezionale, alle acque minerali, di cui siamo ricchissimi, per non parlare di Matera, capitale della cultura.

non avere la volontà di affrontare questi discorsi, cosicché l'unica cosa che resta da fare alle opposizioni - sempre in modo corretto e mai mancando di rispetto a nessuno - è far conoscere con forza quello che succede in quei territori.

se l'unica cosa che aumenta in Basilicata è il numero delle malattie, ci sarà un perché; se 3.000 giovani, su una Regione di 550.000 abitanti, vanno via senza farvi ritorno, ci sarà un perché.

la prima riflessione che mi viene in mente è che forse di queste mozioni di sfiducia oggi potevamo fare anche a meno, con tutto il rispetto che ho per questo strumento democratico che democratico che trova una giusta collocazione nel nostro sistema istituzionale. Ho sentito l'illustrazione delle mozioni di sfiducia, che mi sembrano veramente prive di efficacia, carenti dal punto di vista della strutturazione politica. Mi sembra siano l'ennesimo atto di debolezza delle opposizioni che hanno sfruttato e hanno colto al volo un episodio, un mezzo scivolone

Per noi di Area Popolare si tratta sicuramente di un appuntamento importante per ribadire, con consapevolezza, coscienza e responsabilità, il nostro appoggio a questo Governo, che riteniamo abbia fatto bene e abbia fatto rialzare la nostra Nazione, intraprendendo un cammino, anche se lento, sicuramente virtuoso e positivo. Ribadiamo con fermezza che, all'interno del Governo, una parte da comprimario o da meri *partner* governativi; sicuramente abbiamo inciso con le nostre idee, con la nostra capacità propositiva, con la nostra progettualità nelle riforme che hanno

abbiamo ispirato molte delle riforme, e di questo siamo sicuramente orgogliosi. Abbiamo contribuito a dare una connotazione a questa a questa coalizione, inizialmente formata da diverse anime difficilmente conciliabili sul piano politico,

a Governo di salvezza nazionale, con il presidente Letta e il presidente Berlusconi, a Governo di riforme, che ha capacità di programmazione e ha dato finalmente risposte agli italiani. E di questo siamo assolutamente fieri. Oggi, purtroppo, non si parla molto di politica. Il prossimo appuntamento in cui ci saranno un confronto e anche uno scontro politico è sicuramente quello di ottobre, la riforma costituzionale,

sforzo massimale per convincere gli italiani che noi per due anni, in quest'Aula del Senato e nelle Commissioni, abbiamo lavorato contro gli interessi dell'Italia e degli italiani. Se questo sarà, allora presidente

evidenziato: abbiamo l'esigenza, presidente Renzi, di unificare questa Nazione, che è divisa in due: abbiamo un Nord e un Sud che vanno a trazione completamente diversa. Per unificare la Nazione vanno bene tutte le attenzioni che sono state messe da questo Governo su Bagnoli, sull'ILVA di Taranto e sulla terra dei fuochi, vanno bene le attenzioni poste sugli investimenti produttivi con gli strumenti di finanza agevolata o agevolazioni fiscali. però abbiamo bisogno di un piano infrastrutturale importante e deciso, che metta al primo posto la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Il ponte sullo Stretto di Messina non è un'opera un'opera che unisce due coste: è un'opera che rende funzionale e valorizza la piattaforma siciliana e il crocevia meridionale sul piano logistico. Abbiamo superato, con questo Governo, diversi tabù ideologici veterocomunisti e tutto quello che ha fatto venire il mal di pancia alla sinistra massimalista. Superiamo anche questo tabù veteroambientalista! È un atto politico determinante per contribuire al rilancio del Sud e dare una dimensione europea

sfiduciare questo Governo è diventato un atto dovuto per il Paese, che merita sicuramente di meglio rispetto a una banda di affaristi come voi! Non è normale quello che abbiamo visto fare, in quest'ultimo anno, all'Esecutivo. E mi soffermo solo su quanto è accaduto in materia di Difesa:

Possibile che la posizione dell'Italia in Libia e gli interventi di natura militare, diretti o indiretti che siano, ce li abbia raccontati il «Wall Street Journal»? Grazie a questo giornale i cittadini hanno saputo dell'utilizzo della base militare di Sigonella per far partire droni armati statunitensi verso la Libia. Presidente Renzi, Sigonella si trova in Sicilia, in Italia, e non negli Stati Uniti d'America! Grazie ai giornali italiani, invece, si è saputo dell'invio di agenti speciali italiani in quel Paese in un numero che rivela piuttosto la preparazione a una guerra. Non è normale che nel mistero rimangano tutte le autorizzazioni e proroghe di concessioni agli Stati Uniti e alle forze Nato di uso delle basi militari italiane per attività la cui natura rimane sotto silenzio. Le ricordo, signor Renzi, il MUOS si trova a Niscemi, in Sicilia, in Italia e non negli Stati Uniti d'America. che non abbiamo il diritto, come italiani, di sapere come viene utilizzato il nostro territorio e quale rischio corriamo? Qualcuno ci ha avvertito che nella base dell'aeronautica militare di Pantelleria sempre in Sicilia, in Italia e non negli Stati Uniti d'America, dove abbiamo potuto constatare noi del Movimento 5 Stelle direttamente, attraverso una semplice visita ispettiva - è ospitato un consistente numero di militari americani, la cui presenza e attività sono avvolte nel mistero assoluto. Qualcuno si è preoccupato di avvertirci che degli armamenti nucleari sono detenuti nella base militare di Ghedi nel bresciano, signor Renzi, che si trova in Lombardia, in Italia, e non negli Stati Uniti d'America? Come lei sa, gli americani anche lì la fanno da padroni, nonostante nel nostro Paese siano vietati l'uso e la produzione degli armamenti nucleari. La popolazione è stata informata del rischio che corre? Non è normale stare in una situazione di continua violazione delle leggi e quasi quasi ne andate anche fieri. le dichiarazioni della ministra Pinotti sulla vendita di sistemi d'arma all'Arabia Saudita. Solo per quelle meritava uno sfratto immediatamente esecutivo da via Venti Settembre. Non è normale che la Pinotti, a margine di un convegno, definiva la fornitura di bombe italiane all'Arabia Saudita come "regolare e nel rispetto della legge". Regolare e nel rispetto della legge? Ministra, ma ci sta prendendo in giro? L'Arabia Saudita è un Paese che viola puntualmente i diritti umani, è in conflitto con lo Yemen e molto probabilmente sostiene anche le milizie dell'ISIS. Ma proseguiamo, se questo non vi basta. Non è normale che, appena una procura indaga, spunti di tutto su tutti i dicasteri. In queste settimane inchieste giudiziarie riportate con dovizia di particolari su tutti i *media* hanno scoperchiato il vaso di pandora hanno rilevato senza ragionevoli dubbi, se mai ce ne fossero, quale sia il vero volto di questo Governo, e cioè un agglomerato di lobbisti che, assieme a componenti delle istituzioni, ha messo su un sistema di *do ut des* in grado di assicurare loro vantaggi convergenti. L'inchiesta della procura di Potenza sul filone riguardante alcune concessioni per il porto di Augusta in provincia di Siracusa - in Sicilia, Italia e non negli Stati Uniti d'America, Renzi - è quantomeno scandalosa. abbiamo capito come taluni personaggi hanno amministrato le Forze armate e sperperato denaro pubblico (acquisti, modalità d'uso dei costosi armamenti, interessi perseguiti), nonché il profilo di alcuni alti ufficiali e di una parte dell'*entourage* del ministro Pinotti, un *entourage* a cui non si vuole assolutamente rinunciare, probabilmente perché in linea anche con i suoi di interessi. Infatti non rimuove l'ammiraglio De Giorgi che, in compagnia di altri sinistri personaggi (come Gemelli, il compagno dell'ex Ministro; Valter Pastena - segni, signor Renzi - capo ufficio bilancio della Difesa e consulente del Ministero per lo sviluppo economico, e il facilitatore Nicola Colicchi), risulta indagato ormai per tutti i possibili reati contro la pubblica amministrazione, tra cui associazione a delinquere, traffico d'influenze e abuso d'ufficio. E se il *dossier*

feste sulle navi, aerei utilizzati come taxi anche per le sue dame di compagnia, risorse economiche impiegate per spese pazze come cavalli bianchi, cabine di lusso e quant'altro in dotazione alla Marina di cui ancora oggi, e sottolineo ancora oggi, è capo di stato maggiore. Gruppo M5S)*. E lei, signor Renzi, insieme alla sua ministra Pinotti, se lo tiene lì. Chissà perché siete tanto affezionati a questo personaggio che, tra l'altro, è arrivato anche all'età pensionabile e, anzi, gli volete anche prorogare il ruolo. Cos'altro deve fare quest'uomo per essere ritenuto da voi riprovevole? Tanto mica spende soldi vostri, ma i nostri e sono soldi che spendete per pagare i vostri festini!

Addirittura sembra che abbiate falsato le carte per convincere il Parlamento ad approvare questo megapiano di rinnovo. Sentite colleghi: qui si parla di falsare delle carte. Ci rendiamo conto? Non è normale che ci abbiate presentato documenti parziali e informazioni distorte sulla vera natura e dimensione del programma. Si è parlato di unità navali economiche e a doppio uso, che sarebbero dovute servire per impieghi di soccorso umanitario e protezione civile. E, alla luce di quanto accade in questi giorni nel Canale di Sicilia, dovete mettervi una mano sulla coscienza. Anche i preventivi dei costi sono falsati, perché non è normale che abbiate indicato spese inferiori a quelle che poi avete previsto nei contratti stipulati dopo l'ok del Parlamento.

lobbisti industriali e militari corrotti. Questo non è più un Paese normale e voi avete una grandissima fetta di responsabilità,

non è normale, agli occhi di un «comune cittadino che con il suo lavoro e i suoi (pochi) mezzi cerca, senza alcun contributo pubblico o privato, forse illudendosi, talvolta anche sbagliando, di migliorare la società in cui vive». Presidente Renzi, al suo insediamento la definii la Wanna Marchi della politica. Purtroppo per gli italiani, il tempo ci ha dato ragione. Mi creda - e lo dico senza polemica - lei ci ha stancato.

gli altri partiti sono i primi a essere invece attaccati a quella poltrona, per ovvi motivi. Ma il motivo non è solo questo. Anche se ci fossero i numeri, una sfiducia posta così non cambierebbe nulla, per il semplice fatto che sostituire delle persone con altre, non cambiando i metodi, gli obiettivi e i contenuti, non cambia assolutamente nulla.

Chiediamoci, però, anche perché: spesso c'è stata un'opposizione che, invece di entrare nel merito delle discussioni e, quindi, di proporsi in modo

ora di finirla con slogan a cottimo, con accuse strumentali non provate e infondate, perché non portano a nulla. È di altro che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di cambiare gli obiettivi, la strategia e i metodi, riuscire a capire anche i meriti e le intenzioni degli altri. Questo Governo si è dato delle scadenze e credo sia giusto dargli fiducia e aspettare i risultati entro quelle scadenze, senza anticiparli. E aggiungo, le tante polemiche che sono state fatte, che preferisco di gran lunga un Paese dove i padri diventano famosi per i fatti dei figli ad uno dove i figli diventano famosi per i padri, perché ciò significa che il Paese dà a tutti la possibilità di evolvere e migliorare. Io penso che questo Governo, al di là di tutti gli errori, abbia mostrato una volontà di cambiamento e di fare. C'è poi un altro motivo per cui non voterò la sfiducia: non vedo alternative credibili, non vedo una

è arrivato anche nella legge di stabilità (evidentemente era destino). Quello che ha detto il senatore Malan riempie tutto quello che il nostro Gruppo pensa su detto punto. Una sfiducia al Governo, però, la si presenta anche su molte altre cose. Siccome il tempo è ridotto, il senatore Lucio Malan ha fatto la sua presentazione e io mi dedicherò ad altro.

Lei ci ha parlato del successo dei ricollocamenti. Sappiamo che si parla di qualche centinaio. Adesso, ha un'altra grande idea e un altro grande progetto per l'Europa. Noi sentiamo tante parole, ma non vediamo fatti, neanche relativamente ai migranti. Ma il problema non è soltanto l'immigrazione, naturalmente. L'immigrazione è uno specchietto che rivela che questo Governo

perché si regge sui nostri voti, non su quelli della sinistra, non su quelli del Movimento 5 Stelle: si regge sui voti del centrodestra. È una maggioranza abusiva. Non avrebbe preferito che su quella scheda fosse scritto il suo nome? Allora sì che non sarebbe abusivo; allora sì che sarebbe il Presidente del Consiglio scelto dagli italiani, che invece hanno votato Bersani.

Io non credo sia corretto fare tutto quello che fa, fare il male del Paese e degli italiani con una maggioranza di questo tipo. Sono sicuro che lei sarebbe molto più contento di essere stato eletto, invece lei è stato nominato, a differenza nostra. Non ci illudiamo, anche oggi lei incasserà la fiducia di quest'Aula,

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, componenti del Governo, colleghe e colleghi, nel preparare il mio intervento ho riletto le mozioni di sfiducia; trascorsi alcuni giorni, celebrato - con l'esito noto - il *referendum*, quanto lontane appaiono oggi dalla realtà e dalle esigenze vere del nostro Paese e dei nostri cittadini. Il sapore di strumentalità e di pretestuosità, evidente sin dal primo momento, ha acquistato ulteriore accentuazione. Questo Governo sta lavorando, e bene, per cambiare l'Italia e rilanciare investimenti, economia e occupazione e ci si attarda, come oggi, in una ritualità sterile che nessun contributo positivo dà in tale direzione. Stiamo ai fatti, analizziamoli con il buon senso di manzoniana memoria. È in atto un'indagine giudiziaria da parte della procura della mia città. Mentre lavora, auspicabilmente in tempi rapidi, per accertare la verità e giungere a sentenza, un Ministro del Governo, non solo non indagato ma oggi definito dai medesimi inquirenti parte lesa, strumento inconsapevole, per motivi di opportunità - e io dico giustamente - si dimette. ripeto: non indagato. L'emendamento in discussione, poi, nel merito è giusto, ovvio, sacrosanto, peraltro non eccepito e neppure eccepibile - salvo voler capovolgere la Costituzione - dall'autorità giudiziaria. Esso afferma semplicemente che, se strategica e di pubblica utilità è la realizzazione del Centro oli per estrarre petrolio, tali devono essere anche le infrastrutture di completamento, i collettori per trasportare idrocarburi a Taranto (o qualcuno preferisce che operino autocisterne e autobotti lungo la già insufficiente viabilità del Mezzogiorno?) e le opere per lo stoccaggio nel porto di Taranto. Ciò in totale coerenza con una visione che condivido e che dovrà essere ulteriormente sviluppata nei prossimi anni, in particolare nel Mezzogiorno.

dunque il *gap* aumenta e non diminuisce. Invertire questo *trend* deve essere una sfida ambiziosa per il suo Governo che, come lei, accetta sempre le sfide ambiziose. Non c'è crescita - lo ha detto anche lei di recente - se non riprendono investimenti pubblici e privati (senatore Quagliariello, ce ne fossero di infrastrutture e di investimenti privati); teoria economica antica, se si vuole, ma che non perde mai attualità, oggi a maggior ragione. Una recente ricerca ANCE evidenziava che nel settore si è passati dai 37 miliardi di euro di investimenti del 2004 ai 18 miliardi di euro del 2013. La scommessa, in parte già vinta (la stessa ANCE prevede finalmente un incremento nel 2016), è aumentare la spesa fino al termine della legislatura. Lo si fa attraverso leggi ed emendamenti che sblocchino l'*iter* incrostato di alcune opere (e l'emendamento in discussione va esattamente in questa direzione), e attraverso la legislazione complessiva affinché normi e semplifichi il settore, dia certezza agli operatori: è il caso del codice degli appalti, di recente riformato completamente con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri. Ho letto - e fa un po' sorridere - in una delle mozioni sottoscritte dai colleghi che bisogna introdurre il *débat publique*, come chiesto anche da un disattento Presidente di Regione. Bene, gli uni e gli altri, e per questi ultimi è un po' più grave, non si sono accorti che questo Governo e questo Parlamento lo hanno già fatto a gennaio, approvando la legge delega sul codice, istituto fondamentale per acquisire il consenso propedeutico dei cittadini, ma che funzionerà solo ad una condizione: che poi, dopo avere a lungo dibattuto, una volta che la decisione sia stata presa, l'opera si realizzi e la volontà del Paese, dello Stato in questo caso, venga rispettata. E qui si torna all'emendamento. Troppe volte burocrazia, apparati e politica locale, soprattutto ma non solo al Sud, bloccano opere attraverso veti, o qualche volta peggio, attraverso comportamenti da veri e propri Ghino di Tacco. La legge obiettivo, superata ed abrogata dal nuovo codice, conteneva una previsione positiva, e cioè che il 30 per cento delle opere strategiche dovessero ricadere nel Mezzogiorno. Bene, passando dal programmato al realizzato, questa percentuale è scesa al 10 per cento. Ecco perché bisogna dare allo Stato centrale più forza per superare le pastoie locali. Qualcuno eccepirà - e lo ha fatto con risposta chiara avuta domenica scorsa - che il petrolio non è risorsa strategica, e che dunque non lo sono le infrastrutture ad esso dedicate; altri hanno provato a dipingere questo Governo come disattento sul fronte delle rinnovabili: ancora, in entrambi i casi, strumentalizzazioni e pretesti. Oggi l'Italia produce il 39 per cento della propria energia dalle rinnovabili, e qui - per carità di Patria - non mi soffermo su un altro ricorrente paradosso. Gli stessi che si oppongono alle estrazioni, poi dicono che i parchi eolici

Presidente, quante ironie negli anni scorsi i colleghi stranieri facevano su di noi evidenziando che la Germania produceva energia solare più dell'Italia, il Paese del sole? Oggi non è più così, anche grazie ai passi in avanti nella tecnologia, nell'innovazione e nell'ingegneria delle risorse, fiore all'occhiello del nostro Paese. Ma per quanto tali percentuali possano aumentare, non è di oggi e nemmeno di un domani vicino l'obiettivo del cento per cento di rinnovabili. Dunque, avendo giustamente abbandonato il carbone e non volendo fare il *fracking*, avremo ancora bisogno delle estrazioni petrolifere. Sarebbe suicida, per usare un'espressione di Prodi, non estrarre il petrolio avendolo, e poi comprarlo all'estero. Mi avvio a concludere. Non mi convince l'approccio da leghismo all'incontrario che troppe volte riscontro in giro, anche nella mia Regione: che brutta rappresentazione data qui, caricaturale e falsa, della mia Regione da colleghi senatori lucani.

dire, parafrasando un motto antico: «Il petrolio è mio e lo gestisco io». È profondamente sbagliato. La politica energetica è quanto di più eminentemente nazionale esista

che possono verificarsi quando una piccola comunità e chi la guida si sentano investiti di autorità e potere decisionale assoluti in una materia così delicata. Rimane il tema tutto aperto - l'abbiamo visto anche con il risultato dell'ultimo *referendum* nella mia Regione di vincere la sfida ancora non vinta da venticinque anni - senatore Barozzino, sarà colpa di Renzi se da venticinque anni non riusciamo a vincerla in Basilicata? *(Applausi dal Gruppo PD)*- di come coniugare e tenere insieme estrazioni e crescita economica, sviluppo e occupazione, avendo sempre come pietra miliare la tutela della salute e dell'ambiente

sia approvato in un altro provvedimento e da altro ramo del Parlamento: è la normale dinamica del bicameralismo e stupisce che ve ne lamentiate voi che volete preservarla; mentre noi vogliamo cambiarla, l'abbiamo cambiata e la cambieremo definitivamente con il consenso dei cittadini al *referendum* di autunno. PD)*. Cari colleghi, c'è un'altra cifra di questo Governo, che comprensibilmente oppositori e detrattori non vogliono riconoscere, ma è nei fatti e disconoscere o fingere nei fatti la realtà è esercizio defatigante e, alla fine, inutile: questo Governo, questo Presidente del Consiglio fanno quel che dicono. Nessuno, anche qui dentro, credeva davvero che avremmo riformato questo ramo del Parlamento: lo abbiamo fatto, così come il Governo ha riformato con il *jobs act*, la RAI, le unioni civili, il codice degli appalti, e potrei continuare a lungo. Ha ridato fiducia e capacità di spesa ai ceti più sofferenti

Parlano e parleranno i fatti concreti, non le polemiche strumentali. E i fatti come i numeri sono argomenti testardi e allora, Presidente, vada avanti. Oggi il Senato respingerà la mozione di sfiducia e le darà più forza: la usi come ha fatto sin qui con l'ambizione e la determinazione che sono nella sua natura e vada avanti per governare il Paese e rendere migliore la vita degli italiani. Questo è il senso stesso e il fine ultimo del nostro fare politica. Presidente, concluderò con Seneca che amo quant'altri mai. «La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione». Lei ha talento. Questo è il momento e questa è l'occasione di cambiare l'Italia.

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, nelle oltre due ore di dibattito abbiamo ascoltato toni e considerazioni profondamente diverse. Se dall'una e dall'altra parte si è cercato di onorare un dibattito alto, come quello che riguarda la mozione di sfiducia al Governo portando argomenti ed elementi, ed elementi, in altri interventi si è scaduti nell'insulto e credo che, prima di qualsiasi intervento, debba essere portato a nome mio e del Governo la solidarietà, in particolare modo, a quei giornalisti che sono stati insultati essendo loro privi del potere di querelare i politici che in quest'Aula hanno detto di loro cose semplicemente inenarrabili. Tuttavia, penso che si debba entrare nel merito della discussione e per farlo ho provato a estrapolare cinque punti, molto diversi l'uno dall'altro, che sono stati espressi dalle due mozioni di sfiducia. Li sintetizzo così. C'è innanzitutto una mozione di sfiducia, quella del centrodestra e di Forza Italia,

che doveva fare» e risponderò, per onorare il dibattito, essenzialmente soltanto a questo e cercando di tenere a freno le caratteristiche più legate alle battute e alle polemiche. Secondo punto: c'è un elemento ancora nella mozione di Forza Italia che, accanto alla manifesta incapacità del Governo, pone il problema della moralità politica. È sempre scivoloso il tema della morale, della moralità e del moralismo nella politica, ma accetto la sfida di rispondere nel merito del tema della moralità politica di un Governo che - così viene espresso nella mozione - si regge sul voto di presunti transfughi.

connesse alla vicenda di Potenza. Anche se il senatore Petrocelli, nella sua introduzione, ha evidenziato come per lui il fatto sia squisitamente politico, nella mozione si parla espressamente di alcune questioni legate all'indagine e credo sia mio dovere rispondere nel merito). Il terzo punto, è legato all'indagine. Può questa indagine compromettere la trasparenza - così l'ha definita poi il senatore Mario Mauro nel corso del dibattito - di questo Esecutivo? Il quarto punto investe in pieno la questione energetica e la scelta di quale politica industriale avere, in particolar modo nel Mezzogiorno e in Basilicata, collegata all'estrazione di petrolio e, più in generale, all'inchiesta di cui andiamo di cui andiamo a discutere. Il quinto, infine, è una considerazione di merito sulle modalità del procedimento parlamentare e sul rapporto tra Parlamento, Governo e, soprattutto, magistratura, di cui credo possiamo discutere a lungo, ma in ordine ai quali faccio totalmente mie le considerazioni del senatore Albertini. Concluderò con una considerazione politica sui lavori di quest'Assemblea e sui due anni che ci attendono. Mi permetterete di evitare di soffermarmi su qualsiasi considerazione che è stata estrapolata rispetto all'argomento di discussione da parte di chi ha parlato di altro, come se questa fosse la sede in cui ciascuno può portare un argomento a piacere: ci sono delle mozioni e io affronterò il tema che le mozioni hanno posto alla nostra attenzione. Parto dalla prima considerazione e mi rivolgo, in particolar modo, a lei, signor Presidente, e per suo tramite ai senatori di Forza Italia: al senatore Malan, al senatore Marin e al senatore Paolo Romani nella sua veste di Capogruppo. Questo Governo sarebbe manifestamente incapace di realizzare ciò per il quale è stato chiamato... ciò per il quale ha chiesto il voto di fiducia. Io credo - senatore Romani, mi rivolgo a lei nella sua veste di Capogruppo - che sia legittimo che voi non siate d'accordo sui provvedimenti, ma che sia impossibile - faccio appello alla sua onestà intellettuale - negare che quegli argomenti che erano stati messi al centro dell'azione programmatica sono stati affrontati, con successo dal punto di vista dell'esito parlamentare, da questo Parlamento e da questo Governo. Mi riferisco espressamente alla riforma costituzionale, sulla quale, peraltro, il vostro Gruppo, nelle prime fasi, ha espresso un parere positivo, salvo poi - del tutto legittimamente - cambiare opinione per note vicende indipendenti dal merito della riforma. Mi riferisco alla legge elettorale, su cui è chiaro che questo Parlamento e questo Senato possano avere opinioni diverse, ma che ha visto finalmente l'organo legislativo riappropriarsi di una funzione che la sentenza della Corte costituzionale sostanzialmente gli aveva tolto. Mi riferisco ai provvedimenti sulle tasse, che probabilmente non sono abbastanza per alcuni, che sono sbagliati per altri, ma che hanno visto in rapida successione: l'intervento da 10 miliardi di euro per 10 milioni di italiani attraverso il *bonus* IRPEF di 80 euro; l'intervento

che era un tema storicamente discusso, per anni, nel dibattito parlamentare e anche nelle relazioni tra Confindustria e sindacati. Tutti, in modo unanime, sostenevano la necessità di non gravare l'imprenditore che volesse creare dei posti di lavoro di una sorta di ulteriore gabella, come era stato fatto - devo dire, ad onor del vero - da un'esperienza di centrosinistra e mantenuto, poi, dai Governi di centrodestra. Questo tipo di attività ha portato oggi a provvedimenti legislativi conclusi. È vero, sul tema della riforma costituzionale siamo in attesa del percorso che porterà al *referendum*, e dunque l'ultima parola sarà dei cittadini, come abbiamo avuto modo di dire in più di un'occasione, ma il dato di fatto è che questo Governo aveva degli obblighi verso il Parlamento, sulla base del voto di fiducia nel primo intervento fatto proprio qui, anche con un tono leggermente provocatorio - lo riconosco,

Dunque, si può condividere o meno il merito dei provvedimenti, ma non vi è nessuno in quest'Aula, dall'estrema sinistra all'estrema destra, che possa negare che quei provvedimenti oggi sono diventati legge. Ce ne sono altri naturalmente, il dibattito li ha evidenziati: dalla responsabilità civile dei magistrati alla riforma della pubblica amministrazione, alla buona scuola, su cui vi è un dissenso forte, non soltanto in quest'Aula ma in alcuni casi anche all'interno del Paese - non voglio negarlo

questo Parlamento sta facendo quello che si era impegnato a fare, e questo Governo sta rispettando gli impegni presi con il Parlamento. Si può non essere d'accordo, ma non si può negare questo dato di fatto. «Ma i risultati non arrivano»: così il senatore Marin si è espresso, citando peraltro alcune cifre semplicemente sbagliate; lo dico senza alcuna polemica, anche perché non credo che sia l'oggetto fondamentale della discussione, ma ci tengo che resti agli atti. Il numero degli sbarchi in questo Paese è infatti passato da 23.838 a 25.285: siamo nell'ordine del 4-5 per cento in più. Naturalmente siamo preoccupati per questo, stiamo attenti, ma siamo ben lontani dal 57 per cento; le garantisco, senatore Marin, che c'è una bella differenza tra

un rallentamento delle nuove assunzioni ma, per essere chiari e restare ai dati di oggi e di tre giorni fa, l'INPS riporta due dati molto semplici: il primo è che nel 2015 vi sono stati, al netto delle cessazioni e delle nuove assunzioni, 911.000 contratti a tempo indeterminato in più

quell'incentivo lo abbiamo votato noi; lo abbiamo voluto noi e siamo molto fieri che questo abbia aiutato gli imprenditori ad assumere e che abbia messo oggi delle persone in condizione di lavorare. infatti una delle questioni sulle quali - avrebbe detto il senatore Mancuso - abbiamo trovato un grande accordo all'interno della coalizione che guida questo Paese, e ci dispiace che qualcuno si sia tirato indietro rispetto a questo impegno perché, come lei ha detto, tutto ciò che crea lavoro fa felice l'Italia e gli italiani. Proviamo comunque a immaginare, come ha detto lei, che siamo in presenza di un *flop act*, utilizzando una definizione, di cui peraltro - non voglio deluderla - il *copyright* appartiene al Capigruppo del suo Gruppo alla Camera, come larga parte della mozione, a giudicare delle espressioni che vengono utilizzate. Andiamo a vedere i dati della disoccupazione, cui ella ha fatto riferimento. Non Non parlo delle percentuali, che sono passate dal 13,2 a sotto il 12 per cento - e penso che qualsiasi italiano possa essere contento di questo - ma, guardando i dati INPS, cosicché non possa avere dubbi su questo, dei numeri delle domande di disoccupazione, e non del periodo precedente in cui c'era l'incentivo pieno: parliamo dei dati di disoccupazione del 2016, perché deve restare agli atti su questo singolo punto come sia strumentale l'accusa nei confronti della riforma del mercato del lavoro. Nel febbraio 2016 si sono registrate 105.654 domande di disoccupazione. Sono tantissime, ma sono il 22,7 per cento in meno rispetto al febbraio 2015.

febbraio e marzo, le domande di disoccupazione sono 254.194, ovvero il -28,6 per cento. Lo dico - e termino sui numeri - perché su questo primo punto vi sia la piena consapevolezza che l'accusa che viene mossa a questo Esecutivo di totale e manifesta inadeguatezza, così come scrive la mozione di Forza Italia, può trovare naturalmente riscontro in un dato soggettivo (ciascuno può avere la propria valutazione), ma trova un'evidente e stridente contraddizione con la realtà: in questi due anni abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi dovremo farlo di più, dovremo farlo meglio e con ancora più intensità, ma il primo elemento su cui vorrei rispondervi è essenzialmente questo ed è di merito. Aggiungo (non sia preso come polemica) che se la riforma del mercato del lavoro fosse stata fatta, come ha fatto la Germania di Gerhard Schröder, negli anni tra il 2003 e il 2005, probabilmente le cose sarebbero diverse.

impressionante. Voglio dire al senatore Marin, che ha detto che questo nostro Paese sta aumentando il debito (parlo del debito sul PIL): le ricordo che tra il 2008 e il 2011 - non farà fatica a ricordarsi qual era il Governo che stava governando in quel momento - il debito rispetto al PIL è passato dal 102 al 116 per cento, per poi crescere ulteriormente - perché mi piace ricordarlo - tra il 2011 e il 2014, dal 116 al 132 Questi sono i numeri e i fatti. Il resto è utile per una comunicazione esterna, alla quale poi verrò nella conclusione finale. Secondo punto: si parla di moralità politica e la moralità politica si interpreta sostanzialmente nel dire che - la sintetizzo così e nel corso della discussione avrete modo, eventualmente, di modificare o precisare il mio pensiero - non si può governare governare un Paese senza un mandato diretto o appoggiandosi a un consenso parlamentare che non è figlio della diretta candidatura. E su questo punto naturalmente in ballo non tanto la moralità politica, quanto, io credo, la Costituzione italiana e le regole del gioco parlamentare. Credo che i custodi e difensori della Costituzione o lo sono sempre o non possono esserlo a giorni alterni. Tra qualche mese (lo avete ricordato tutti) andremo ad un grande dibattito sulla Costituzione dove una parte di voi difenderà la Costituzione per com'è, sostenendo con forza il rischio di un accentramento di poteri nel Presidente del Consiglio. Evito di riprendere qui una discussione già fatta sia al Senato che alla Camera, e cioè che questo argomento è manifestamente infondato perché non si cambiano i poteri del Presidente del Consiglio, a differenza della riforma costituzionale approvata dal Parlamento e poi bocciata dai cittadini nel 2006. se vogliamo prendere sul serio questa critica, dobbiamo essere coerenti fino in fondo: il sistema che voi difendete (e che peraltro rimane in vigore), è quello che prevede la centralità parlamentare e la centralità parlamentare, per effetto dell'articolo 67 dell'articolo 67 della Costituzione e del divieto di mandato imperativo, permette ai deputati e ai senatori di fare le proprie valutazioni. O questo vale sempre, o non vale mai. senatore Malan ha espresso nel suo intervento un riferimento al 2011. Senatore Malan, lei ha detto che il 2011 è stato l'ultimo anno in cui il Governo aveva la piena legittimità. Le segnalo che, a fronte di una frattura nello schieramento di cui lei fa parte e di una divisione profonda effettuatasi nel dicembre del 2010, quel Governo già nel 2011 si basava sul consenso di deputati e senatori, che lei potrebbe definire transfughi ma che nel passaggio parlamentare, del tutto legittimo costituzionalmente per rispondere all'accusa di immoralità politica, passarono dal centrosinistra al centrodestra, sostenendo il Governo Berlusconi. *(Applausi dai

Presidente, io continuo tranquillamente perché avendo fatto un voto di tranquillità e serenità tornerò sui singoli punti anche qualora la maleducazione dovesse continuare ad interrompere, offrendo un pessimo servizio agli studenti che pensano che il Senato sia un luogo di bellezza e di democrazia. *(Applausi dai Senatore Paolo Romani, ma come fate a scrivere in una mozione che esiste un problema di moralità politica quando lo schema di Governo che oggi viene replicato, in modo diverso, è stato alla base del vostro sostegno all'esperienza del Governo Letta, che è venuta meno non in virtù di un giudizio dell'Esecutivo guidato dal mio predecessore ma di una dinamica processuale legata al vostro capo di partito. Il vostro cambiamento di giudizio rispetto al Governo Letta non è derivato da un giudizio politico sul Governo Letta ma dal fatto che avete scelto di togliergli la fiducia in virtù di una vicenda processuale del presidente Berlusconi. Come potete contestare agli amici di NCD prima e poi agli amici di A-LA, che hanno sostenuto il percorso delle riforme costituzionali che voi stessi avevate immaginato, di rimanere semplicemente fedeli ad un patto al quale anche voi vi eravate legati e dal quale siete venuti meno non per esigenze di moralità politica ma per correttissime valutazioni di opportunità?

il tema della giustizia. Io sono per la giustizia sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni.

e invitiamo la magistratura ad andare a sentenza, noi non stiamo accusando la magistratura: noi stiamo rispettando la Costituzione italiana sulla quale abbiamo giurato ed è bene che il Parlamento sia consapevole di questa posizione del Governo. Questo Paese ha conosciuto figure di giudici eroi che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione e contro l'illegalità. Ma questo Paese ha conosciuto anche negli ultimi venticinque anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo. Un avviso di garanzia, strumento processuale a tutela dell'indagato, è stato per oltre vent'anni una sentenza mediatica definitiva. Vite di persone perbene, sviluppo economico*. ...sono state distrutte mentre i delinquenti avevano il loro guadagno nell'atteggiamento demagogico e populista di chi faceva di tutta l'erba un fascio. E oggi io dico, davanti a quest'Aula, che l'avviso di garanzia non è mai una condanna e dico all'assessore dei 5 Stelle di Livorno che noi non chiederemo le sue dimissioni perché è stato indagato perché crediamo nella Costituzione e crediamo nei processi che si fanno nelle aule. Rivendico in quest'Aula, guardando negli occhi i cultori del giustizialismo a senso unico, che chi è colpevole e chi non è colpevole viene deciso seguendo un *iter* processuale, con le garanzie che vengono da un Paese che ha dato i natali a Beccaria. Contano i codici delle leggi non i codici di un *software* per decidere chi è colpevole.

alla separazione dei poteri. Lo dico al senatore Quagliariello, del quale mi ha colpito la clamorosa superficialità, che da lui non mi aspettavo,

magistratura di Potenza possano finalmente essere emanate in primo, in secondo e in terzo grado. Lo abbiamo fatto in tempi non sospetti, quando uno di noi, che ha parlato oggi in quest'Aula e a cui va la mia gratitudine, il senatore Margiotta ha avuto un comportamento di una civiltà straordinaria, dimettendosi dal suo Gruppo parlamentare, per non infangare, alla luce di quello che stava accadendo nel dibattito esterno. Il senatore Margiotta, attesa la sentenza, è stato giudicato innocente. Finché c'è questa Carta costituzionale - e su questo punto la difenderemo con le unghie e con i denti caro senatore Quagliariello, le sentenze sono quelle che passano in giudicato. Non è sfortuna aver detto che non vanno mai a sentenza; le indagini del 2001, le indagini del 2004 e le indagini del 2008 non avranno una conclusione con una sentenza passata in giudicato. CAPPELLETTI *(M5S)*. Vanno tutte perché io, da cittadino, penso che quando un magistrato è messo nelle condizioni di lavorare, deve essere aiutato e accompagnato dal sostegno e non dalle critiche. Quando però non si arriva a sentenza e si immagina semplicemente di condannare le persone sulla base delle comunicazioni date ai giornali, in quel preciso momento mi ergo dalla parte della giustizia,

Preciso, per la superficialità con cui sono intervenuti alcuni senatori, che non voglio neanche citare, che non vi è alcuna ipotesi di corruzione che riguarda questo Governo. Credo che l'unica ipotesi di procedimento penale che nascerà da questa vicenda sarà quella su cui vi chiameremo a rispondere della diffamazione nei confronti del Partito Democratico e su cui spero che voi cittadini rinuncerete all'immunità parlamentari *(Applausi Lì vedremo chi sarà condannato e chi no. Ma voglio dire una cosa: ci sono 400 persone che, da domani, saranno in cassa integrazione e sono i dipendenti dell'ENI di Viggiano. *(**Commenti dal Gruppo Quando avranno finito con le loro urla, torneremo alla dura verità dei fatti e sarà per loro un piacere passare alla concretezza, dopo tante discussioni fatte per chi sta fuori da qui.

e voglio dire a qualche senatore dell'area che, se non ci fosse stata una sacrosanta battaglia di qualcuno di noi a difesa di Fiat Chrysler, oggi ce ne sarebbero molte di più a Melfi. E non può bastare una battaglia ideologica per spiegare che, se c'è un futuro per questo Paese, è un futuro industriale, non un futuro da Disneyland dei servizi, e mi piacerà vedere come voterete voi su questi passaggi della mozione. voglio dirvi una cosa: i giudici devono parlare con le sentenze e noi li aspetteremo, li incoraggeremo e saremo dalla loro parte. Ma le sentenze devono arrivare presto, perché noi vogliamo sapere chi è il responsabile, vogliamo sapere chi è il colpevole, vogliamo sapere chi è che ruba, perché la differenza che c'è tra chi dice che rubano tutti e chi dice "datemi i nomi" è esattamente la stessa differenza che c'è tra quelli che non vogliono nessun colpevole, sparando

Vedete, è la stessa differenza che c'è tra interpretare la politica come servizio, come grande servizio, e interpretare la politica come grande *server*. *(Ilarità)*. È una grande differenza, ma è una differenza che però potranno capire soltanto con il tempo, perché prenderla tutta insieme potrebbe essere difficile. Vi è un quarto punto, che riguarda l'energia e le politiche industriali. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente del Senato. Il dibattito sulle mozioni ha toccato soltanto *en passant* la questione di quale politica industriale avere per il Mezzogiorno. Io vorrei ribadire qui, in questa sede, qual è la politica energetica e industriale di questo Governo. Oggi che il passaggio referendario si è concluso e oggi che sembra venir meno l'attenzione su questi temi, proprio oggi è necessario dare nuova luce alle questioni dello sviluppo energetico ambientale e della politica industriale di questo Paese. Per questi motivi tra due giorni sarò a New York, con gli altri Capi di Stato e di Governo, a firmare l'impegno vincolante della Conferenza di Parigi. Noi pensiamo che le centrali a carbone

la riconversione da olio a carbone, abbiamo messo lo stop. Con ENEL blocchiamo pertanto cinque centrali in questa legislatura, senza perdere un posto di lavoro, perché ENEL si è impegnata a riqualificare tutte le lavoratrici e i lavoratori di quelle realtà. Siamo *leader* nel settore delle rinnovabili, e vorrei essere chiaro su questo. Il sistema degli incentivi,

(grande argomento, di cui potremmo discutere a lungo) e sono oggi sempre meno necessari, perché si sta affermando l'idea delle energie alternative rinnovabili come valore profondo, che funziona in molti casi anche senza incentivi, cioè senza pesare sulla bilancia dei pagamenti e soprattutto sulla bolletta dei cittadini. *(Commenti della senatrice spuntino sotto il cavolo non è propriamente veritiera; gli incentivi vengono pagati dagli italiani con una bolletta energetica che è tendenzialmente più alta di quella degli altri Paesi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Dunque, sulle rinnovabili abbiamo raggiunto gli obiettivi per il 2020, saremo in grado di essere i *leader* nel percorso verso gli obiettivi per il 2030 e andiamo avanti con grande determinazione e convinzione. Abbiamo il tema dell'efficientamento degli immobili. Chi ha fatto il sindaco sa che una delle più belle esperienze che gli possano capitare non è soltanto quella di collegare con un collettore le fogne a un depuratore. Infatti, si parla tanto di ambiente, ma poi ci si dimentica che il vero modo per difendere il nostro mare è quello di creare le condizioni per fare i depuratori e - come sappiamo molto bene noi che abbiamo fatto i sindaci - per mettere le fogne in condizione di essere collegate a un depuratore. *(Applausi dal c'è il tema dell'efficientamento degli immobili. È inutile continuare a fare discussioni*spot*, se tu non metti in campo una politica per rendere più efficiente dal punto di vista energetico gli immobili. Una delle esperienze più belle, da sindaco, è stata quella dell'edilizia residenziale popolare (ERP), fatta con i livelli di massima efficienza energetica. Ci sono ex sindaci, in quest'Assemblea, che hanno fatto esperienze molto interessanti. poi il tema cruciale delle colonnine elettriche per la mobilità elettrica privata. Noi abbiamo circa 2.000 colonnine elettriche; se non arriviamo a 20.000, non siamo credibili. C'è il tema del rinnovo totale dei mezzi pubblici.

Pertanto, se vogliamo affermare la necessità di un cambiamento di paradigma in questo settore, occorre mettere da parte la cultura anti-industriale che ha permeato una parte della classe dirigente di questo Paese, soprattutto del Mezzogiorno, e che ha visto distruggere, nel corso degli anni, alcune realtà straordinariamente forti ed efficaci.

economica. Questo è il grande tema che, come Governo, stiamo cercando di perseguire. Ed è il quarto argomento, talvolta assente da questo dibattito, preso probabilmente

come è accaduto purtroppo a tanti giornalisti e a tanti politici nei *talk show*, una tesi che non sta né in cielo né in terra. Questo emendamento è stato discusso proprio al Senato. E mi dispiace dovere essere io a dirglielo. Non entro nel merito della rivendicazione di quell'emendamento. Non lo faccio perché vi sono interviste pubbliche mie, fatte tra il mese di giugno e quello di settembre, in cui spiego la strategicità di Tempa Rossa, che poi si può non condividere. Riconosco in questo caso al Movimento 5 Stelle di essere sempre stato contrario nel merito. Ma con la stessa franchezza, voi dovete riconoscere a noi che abbiamo sempre chiesto che questo emendamento fosse portato. Lo abbiamo detto in tutte le sedi. Qual è il punto? Sì, è vero che esso è arrivato alla conclusione dei lavori parlamentari della Camera, ma questo emendamento è stato discusso in sede di Commissione. E le dirò di più, senatore Malan: a sua insaputa è stato anche subemendato.

Il fatto che abbiate votato contro è assolutamente legittimo. Nessuno di noi vuole mettere in discussione che abbiate votato contro. Ma il fatto che se ne sia discusso e che sia stato approfondito in sede di Commissione

Io rivendico qui, in quest'Assemblea, gli interventi che il Governo fa allo scopo di sbloccare le opere pubbliche e private.

che noi abbiamo inteso sbloccare, come abbiamo inteso sbloccare l'Expo; come rivendichiamo il commissariamento del Mose; come abbiamo inteso fare per la Variante di Valico, per la Salerno-Reggio Calabria e per il Quadrilatero. Pensiamo infatti che questo Paese abbia bisogno di sbloccare gli investimenti.

dei nostri Comuni, dai nostri amministratori e in questa sede li rivendichiamo. Se è un peccato, o se volete un reato (anzi, se è un peccato, sul reato ci torneremo tra un attimo); se considerate un peccato cercare di sbloccare l'Italia, accusateci di questo peccato. Se lo considerate un reato, controllate il codice penale, perché il reato non c'è.

questo significa poter governare degli interessi. Inoltre, rispondiamo di quello che facciamo in piena libertà e a viso aperto, utilizzando un'espressione peraltro molto cara a chi di noi ama Dante e Farinata. L'altro giorno al Salone internazionale del mobile di Milano ho incontrato il presidente della Snaidero. Vorrei fare una confessione pubblica in Parlamento. Noi abbiamo presentato la legge di stabilità

Questo è l'esercizio democratico: prendere le considerazioni che vengono dal mondo fuori di qui, valutarle in scienza e coscienza sulla base dell'interesse pubblico ed esprimere una valutazione. Questo significa dar retta alle *lobby*? Noi siamo il Governo che ha messo l'ANAC in condizione di funzionare. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Voi siete il Parlamento che ha aumentato le pene sulla corruzione, che ha introdotto i reati ambientali, che ha fatto interventi che definire figli delle *lobby* non riesce neanche a chi vive nell'Iperuranio. Questi sono i cinque temi su cui vi dovevo una risposta di merito puntuale, avendo ascoltato il dibatto e avendo letto le mozioni. Certo, ho perso un po' di stimolo all'inizio del dibattito. l'onorevole Di Maio e l'eurodeputato Salvini avevano spiegato sui giornali e nei *talk show* che questa mozione sarebbe passata, quindi sono arrivato con un misto di tremore e anche d'interesse, ma il senatore Centinaio ha subito spento la mia emozione intervenendo in Assemblea dicendo: tranquilli, questa non passa; sarà la prossima, quella del *referendum*. Siamo ormai abituati a sentirci dire che non sarà questa ma la prossima. Aspetteremo pazientemente la prossima, ma nel frattempo vorrei farvi una proposta. Per l'ennesima volta provate a mandarci a casa non convinti neanche voi di farlo, ma evidentemente per due ragioni: o perché vi piace perdere (ma non credo perché non piace a nessuno), o perché pensate di giocare così la vostra attività politica, utilizzando il Senato come la cassa di risonanza per ciò che sta fuori, utilizzando la mozione di sfiducia, non come uno strumento parlamentare,

Questo atteggiamento è del tutto legittimo e non tocca a me chiedervi di cambiarlo, perché credo nel rispetto e nel gioco democratico. Penso però di dovervi dire con estrema franchezza, per la stima e il rispetto che porto al Presidente del Senato e a tutti voi, che i *talk*, i *media,* i *social* non sono l'Italia. Spero che ve ne siate accorti con l'ultimo *referendum*; spero che ve ne siate accorti in ogni passaggio: non sono i sondaggi che vengono più o meno agitati, prima dell'uso. Noi politici troppo spesso viviamo in una grande, gigantesca bolla di autoreferenzialità. ai lavori (molto spesso gli addetti ai livori), immaginano che abbiano grande interesse certi temi, mentre le persone che sono a casa in questo momento

È nato così un *referendum* che è in entrambe le mozioni la conclusione della mozione. Senatore Paolo Romani, che questo sia stato fatto da altri si vede, perché la conclusione della mozione di Forza Italia dice l'esatto contrario di quello che lei ha mirabilmente spiegato in un'intervista su «Il Foglio»; evidentemente ha preso la cartellina della mozione della Camera. La prossima volta siamo più tranquilli se prende la sua. Nasce così la richiesta di sfiducia, finalizzata soltanto ad avere eco fuori di qui, e nasce così un discorso in quest'Assemblea che fa l'occhiolino a chi sta fuori, ma che non guarda alla sostanza del problema.

«la politica è altrove, noi vi aspetteremo là». Io credo che sia la stessa cosa che dobbiamo dire oggi. La politica è rispettare chi governa, non urlare costantemente, facendo un'opposizione costruttiva, preparandosi a governare la volta dopo, rispettandosi - cosa che abbiamo cercato di fare con il patto del Nazareno - e non delegittimandosi vicendevolmente. L'Italia è altrove, la politica è altrove; quando avrete finito con le vostre sceneggiate televisive, noi vi aspetteremo là.

Numeri, questi, elaborati dai Medici per l'ambiente dell'ISDE. Corleto si trova a quattro chilometri in linea d'aria dal centro di Tempa Rossa, finito nell'occhio del ciclone giudiziario e politico.

Anche il registro dei tumori, che dovrebbe essere una fonte importante di dati, per quanto riguarda la Basilicata, non è stato ancora accreditato: perché tutto questo? secondo punto, che ritengo più importante: il *blitz* dell'antimafia sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pozzi petroliferi dell'ENI e trasportati all'impianto di smaltimento della Tecnoparco di Pisticci, ha visto oltre trenta avvisi di garanzia. Il senatore lucano del Movimento 5 Stelle, Vito Rosario Petrocelli, oggi era molto arrabbiato; promise molti mesi fa una Norimberga ambientale in Basilicata. Invece, in occasione della visita della Commissione industria del Senato, agli impianti dell'ENI e della Tecnoparco, nel giugno del 2014, affermò che: «ENI ci rassicura sulla reiniezione petrolifera», «parlare con ENI è stato positivo, la posizione del Movimento in materia è chiara». Avrei bisogno di capire meglio che cosa è chiaro, visto che in un comunicato di Giorgio Santoriello, sul senatore grillino, si legge: «Pesantissimi i suoi silenzi e le mancate denunce postume ai sopralluoghi suddetti, che sanno di passerelle nonostante la qualifica di geologo del senatore stesso, invece nulla, a testa bassa ed in silenzio come sempre». La testa la alza solo qui dentro. In Tecnoparco Valbasento lavora, come responsabile ambiente, sicurezza e qualità, la dottoressa in chimica Maria Teresa Adamo, moglie del senatore Petrocelli. E conclude: non è un evidente conflitto di interessi del senatore Vito Rosario Petrocelli? Vengo al terzo ed ultimo punto: il tenente della polizia provinciale di Potenza, Giuseppe Di Bello, e i radicali lucani, nel gennaio del 2010, autofinanziarono analisi indipendenti per fare luce sullo stato di inquinamento di alcuni invasi in Basilicata. Per questo, il tenente Di Bello subì una condanna in primo e secondo grado, per essere poi assolto da tutte le accuse in Cassazione. Ma non fu assolto da Grillo e Casaleggio. Forte della sua celebrità sbaraglia tutti gli altri candidati alle regionali *online* del Movimento 5 Stelle. A questo punto afferma di essere stato contattato prima dal senatore Petrocelli e poi dallo stesso Grillo, che, in modo scortese, lo avverte che deve fare un passo indietro. «Lì mi risveglio dal sogno - dice Di Bello - capisco che il Movimento 5 Stelle è solo un prodotto di *marketing*, non serve a cambiare il Paese». chi si occupa della tutela della salute dei cittadini della Basilicata se maggioranza da un lato e opposizione dall'altro non sembrano poi così lontane nel modo di operare? Spero non solo noi dell'ISDE. Per il momento mi ritengo soddisfatto delle dimissioni del ministro Guidi e mi auguro che il Governo approfitti di questo ennesimo scandalo per dimostrare che il suo impegno contro la corruzione non è solo a parole ma anche nei fatti. Per questo noi dell'Italia dei Valori diciamo no a queste mozioni di sfiducia.

e che lei ha testimoniato così bene nella regolare discussione. Come vede però, dal Governo non abbiamo lo stesso trattamento. Vorrei tranquillizzare i signori del Governo: questa non è un'aula di tribunale. Qui non c'è nulla di cui avere paura. Abbiamo già abbastanza da fare nell'affrontare i tanti nodi politici che scaturiscono anche dalle vicende giudiziarie da non avere tempo ed energie per sovrapporci all'attività della magistratura. Io valuto e giudico la responsabilità politica legata all'opportunità o meno di azioni e proposte e non altro. Certo, tranquillizzo il presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha potuto notare che, all'interno di questa mozione di sfiducia, anche solo i toni, che noi non abbiamo condiviso, ma che per il valore supremo dell'unità del centrodestra abbiamo accettato, gettano nel ridicolo questa azione e, soprattutto, fanno rivivere nei sorrisi di Paolo Romani quel patto del Nazareno che c'è e lotta con lei, signor Presidente del Consiglio, che se ne è andato.

può essere garantita da un carsico e strisciante patto del Nazareno, che è ancora uno degli elementi drammatici che inficia e ammorba l'attività di opposizione seria e responsabile, come quella svolta dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti, che proprio per quella vicenda uscì da Forza Italia, e dai colleghi della Lega che, insieme,

non siamo qui ad accettare da lei patenti di solidarietà o di rispetto nei confronti dei giornalisti, perché lei è stato fatto oggetto di attacchi da parte di autorevolissimi giornalisti, che che denunciano il tentativo da parte sua di imbavagliare importanti trasmissioni televisive per anestetizzare il dibattito pubblico, come ha fatto così bene sul *referendum* delle trivelle. Ma siamo qui per ripercorrere brevemente i punti più importanti della cosiddetta vicenda Tempa Rossa, che vedono pericolosamente intrecciarsi questioni di rilevanza nazionale. Su questo lei ha ragione, Presidente del Consiglio, che non c'è più; se poi ora va via anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento siamo proprio alla frutta, per un Governo che, come vede, non riesce a misurarsi nemmeno con il suo Parlamento, figuriamoci con tutti gli altri. È, infatti, di rilevanza nazionale - e ha ragione il presidente Renzi - la politica energetica del sistema-Paese, ma lo sono anche le attività delle *lobby* e queste vicende personali che si intrecciano pesantemente Grazie a tutte un soggetto privato straniero e non certo pubblico o italiano come, ad esempio, è l'ENI. Ma quelle riunioni erano finalizzate evidentemente a studiare un percorso legislativo che agevolasse l'attività estrattiva dell'azienda francese, che ovviamente si muoveva sulla base di logiche di profitto, in qualche caso anche speculative, perché risparmiare i soldi sulla messa in sicurezza di quei pozzi e sul *decommissioning*, come viene definito, significa speculazione, pur assolvendo agli oneri di legge riguardanti le *royalty* sui materiali da estrarre. Questo sta molto a cuore ai cittadini della Basilicata, perché da questo dipende anche una parte del loro Il Governo decide di estendere la qualificazione di opere strategiche anche a quelle necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali e strumentali, anche lontano dal giacimento, sottoponendole al regime di autorizzazione unica per opere di tipo strategico. Ma la strategia dello sviluppo della politica energetica ha al suo centro i siti in cui si svolge; le opere di trasporto e la logistica non è detto che lo siano altrettanto. Ma a bloccare ogni opposizione da parte degli enti locali si è frapposto il secondo comma dell'emendamento incriminato; lo sblocca Italia, infatti, prevede che, in quanto strategiche, anche su quelle opere la decisione finale spetti al Governo. Il via libera arriva di 19 dicembre 2015, quattro mesi fa, quindi. Chi firma quel testo? Lo firma il ministro Guidi, ma, successivamente, si interviene con un subemendamento del relatore. Ecco dove Renzi può ricordare che il Senato ha lavorato su quel testo: lo conosceva, perché è il relatore che modifica addirittura la condizione del parere vincolante del Ministro dell'ambiente con un semplice «sentito»;

Questo è proprio lo stile del Presidente del Consiglio, che poi è anche il segretario del Partito Democratico e che oggi è anche il Ministro dello sviluppo economico: si bypassano persino i Ministeri competenti per materia e si porta ogni decisione a Palazzo Chigi. Pochi che gestiscono tutto e, come si è visto, non sempre in trasparenza. Il punto chiave della vicenda, almeno per quanto riguarda il Parlamento (quello che sta a cuore a noi), è proprio quell'*iter* legislativo. Grazie a tutte legge elettorale che alle 6,40 del mattino doveva essere incardinata, ma solo dopo avere votato una legge di stabilità che veniva approvata da una maggioranza con la fiducia su un testo, un maxiemendamento, che - tutti ricordiamo - gettò nell'imbarazzo il vice ministro Morando per paragrafi che non corrispondevano al testo, numeri sbagliati, pagine volanti. Sembrava un film comico, e invece era una notte tragica nella quale, per la furbata dell'incardinamento di una legge elettorale Grazie a tutte

momento, ma sono certa ci sarà), autorevole componente di questa maggioranza, che aveva tutto il titolo a firmare quel testo. Tutto ciò, a nostro avviso, getta un'ombra inquietante sul Governo in relazione a quel dovere istituzionale di cura e salvaguardia dell'interesse pubblico, di tutela del territorio e dello sviluppo nazionale, che è ciò che deve stare più a cuore

aver costretto il ministro Guidi alle dimissioni, avoca a sé la paternità di quell'emendamento, dicendo che era suo. A questo punto la logica dice: se si è dovuta dimettere il ministro Guidi, forse è quanto mai opportuno che si dimetta il *premier* Renzi, se proprio era suo quel testo. Senza in alcun modo confondere il ruolo del Parlamento con le indagini in corso, a noi appare necessario verificare la filiera delle decisioni: questo è un nostro preciso dovere. Ecco perché il Gruppo dei Conservatori Riformisti, su proposta del senatore Di Maggio, ritiene necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare che faccia luce proprio su quella filiera delle decisioni, a garanzia dell'interesse pubblico supremo e a garanzia di quel punto di equilibrio tra lo sviluppo che noi dobbiamo percorrere e rincorrere, tra politica energetica e tutela della salute dei cittadini Signor Presidente, tutta questa vicenda, ha prodotto almeno l'accelerazione della discussione attorno alla proposta di legge che regoli finalmente la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, però attenzione a non rendere la toppa peggiore del buco. La commistione di vicende giudiziarie sotto la pressione mediatica e il dibattito sul *referendum* rischiano di inquinare un sereno dibattito sul tema. Presidente - ha visto contrapposti, da un lato, la difesa dell'ambiente, dall'altro, la tutela di una pseudo politica energetica che non c'è. Non c'è nelle azioni di Governo; non c'è in quel DEF che viene valutato così negativamente da tutti gli osservatori internazionali (ma positivamente solo dagli amici del Presidente del Consiglio); non c'è nell'azione attuale del Governo e soprattutto non c'è nel futuro del nostro Paese. Questo è il motivo, il vero motivo per cui vale la pena di votare questa mozione di sfiducia.

L'interlocutore in questo momento è il Senato della Repubblica, composto da senatori eletti dai cittadini italiani che non meritano il «pippone» di quaranta minuti che ci siamo sorbiti da parte del dottor Renzi,

C'è una mozione di sfiducia importante, promossa da buona parte del Senato, sicuramente non la maggioranza perché non abbiamo la maggioranza (ne abbiamo già parlato), però penso che il rispetto di cui ha parlato il dottor Renzi poc'anzi sia doveroso. Lo stesso rispetto che il dottor Renzi non ha avuto, se vi ricordate, durante il primo passaggio della riforma costituzionale, quando in quest'Aula si discuteva la soppressione o la finta soppressione del Senato della Repubblica e lui era bello bello a guardarsi le partite di calcio; lo stesso rispetto che lui non ha avuto nelle interviste, quando, a proposito dei senatori, in modo in modo altezzoso, ha sempre parlato di persone che erano presenti in Aula o partecipavano al dibattito Parlamentare solamente per quindi che quello che deve essere ricordato a questo Presidente del Consiglio è che un po' di rispetto nei confronti dell'interlocutore è doveroso. Ma, ahimè, parliamo a questo Presidente del Consiglio che non esiste. La prossima volta porterò un cartonato del Presidente del Consiglio quando lui deciderà di andare via metteremo lì un finto Presidente del Consiglio, un bambolotto, un cicciobello di turno, così almeno sembrerà che qualcuno ci ascolti.

non è lo stesso dato rispetto all'anno precedente. Ahimè, il dottor Renzi è purtroppo un po' disinformato: anche quando parliamo di lavoro sappiamo benissimo che nulla o molto poco è stato fatto per far crescere il tasso di occupazione nel nostro Paese.

che purtroppo sono state approvate, che piacciono al dottor Renzi e a qualche suo amico e servono a riempire qualche pagina di giornale e a mandare i parlamentari del Partito Democratico in quei *talk show* tanto osteggiati dal nostro presidente Renzi. Ricordiamo al presidente Renzi che anche il tasso di disoccupazione giovanile è ancora sopra il 40 per cento. Ricordo al Presidente del Consiglio quando il Partito Democratico, durante il Governo Berlusconi, uscì con una serie di manifesti in tutta Italia con su scritto: «Disoccupazione giovanile al 29 per cento: Berlusconi dimettiti». E qui cosa dobbiamo dire? «Disoccupazione giovanile al 40 per cento: Renzi sparati»? No! Gli diciamo: vattene a casa che forse è meglio, per tutti quei giovani che sono qui ad aspettare la sua transumanza. Il dottor Renzi ci ha raccontato - e lo abbiamo ascoltato con attenzione, contrariamente a lui, che con i suoi visini, quando gli stavamo parlando, sembrava pensare a tutt'altro - un mondo fantastico, un'Italia che vede lui: un'Italia che riparte, un'Italia che esce dal tunnel, un'Italia cui gli italiani beneficiano di tutte queste bellissime riforme, riformette e riformone che questo Presidente del Consiglio ed il suo Esecutivo hanno fatto per loro.

Ricordiamo al dottor Renzi e ai suoi amici cosa ne pensano gli insegnanti di questo mondo fantastico di cui lui parla, di quel concorso farlocco che sta ammazzando la scuola e gli insegnanti precari. *(Applausi della senatrice Mussini).* Ricordiamo al dottor Renzi e ai suoi amici cosa ne pensano le Forze dell'ordine, quotidianamente davanti a Montecitorio a protestare.

pensano i pensionati di questa bellissima Italia che ci ha raccontato il signor Renzi: beneficiano delle sue riforme, beneficiano dei soldi che la signora Fornero gli ha rubato e che lui non non vuole restituire loro? Ricordiamo e chiediamoci cosa pensano i giovani costretti ad emigrare sempre di più. Esportiamo menti e importiamo dementi che massacrano il nostro Paese. Chiediamoci, in questa Italia stupenda e bellissima, cosa pensano i truffati dalle banche che stanno ancora aspettando quei soldi che lui gli aveva promesso, e ogni settimana dice che, sì, arriveranno, arriveranno. Eh! Arriveranno, Pensiamo a cosa pensano i commercianti ammazzati dalle tasse, ogni anno sempre più care, vengono abbassate saracinesche e di conseguenza sempre più famiglie allo sbando e sempre più famiglie in giro. Pensiamo a cosa pensano gli enti locali: lui arriva dagli enti locali e teoricamente avrebbe dovuto tutelare i Comuni e le Regioni e invece no: tagli su tagli su tagli, con i sindaci che sono obbligati, grazie ai suoi tagli, ad aumentare le tasse locali e diventare un po' come lo sceriffo di Nottingham. Lui fa il fenomeno promettendo gli 80 euro a destra e a sinistra, tra un po' li prometterà veramente anche se hai un gattino, un cagnolino o un cavallino, mentre i Comuni e i sindaci sono sempre più allo sbando. Pensiamo a cosa pensano i malati che subiscono i tagli alla sanità. Lui continua a dire di no, tutti gli indicatori ci dicono di sì. Mettetevi d'accordo. Il problema è che le Regioni continuano a subire tagli e di conseguenza bisogna tagliare sulla sanità, ma chi se ne frega, viviamo in una Italia stupenda e bella, l'Italia del mulino bianco del Presidente del Consiglio! Pensiamo a cosa pensano i parenti di tutte quelle vittime che grazie al suo svuota carceri, agli svuota carceri che sta facendo il Presidente del Consiglio insieme ai suoi amici, subiscono l'umiliazione, oltre ad aver subito un torto, di vedere i cosiddetti Caino fuori, in giro a festeggiare.

noi non abbiamo mai cambiato idea, contrariamente ad altri, noi non abbiamo appoggiato Monti, contrariamente ad altri, noi non abbiamo appoggiato Letta, contrariamente ad altri, e noi non sosterremo mai - ahimè per lui - un Governo presieduto da questo Presidente del Consiglio. Concludo, signor Presidente, dicendo che logicamente noi voteremo Grazie a tutte all'assente di turno che non è ancora arrivato (lo ripeto per chi ci ascolta che non è ancora arrivato): questo Governo vede la luce in fondo al tunnel. Spero che non sia il tunnel del Gottardo, visto e considerato che in geografia

Non me ne dolgo, per il fatto che non siano qui ad ascoltarci: la giornata è lunga e l'orario è tale che bisogna anche andare sui telegiornali. Quindi, vado subito al tema dell'intervento. e rappresentanti del Governo, forse il *referendum* non è un dovere popolare e ce lo hanno ricordato personaggi molto augusti e importanti della vita politica

il voto di fiducia è stato pensato dai Padri costituenti - e il professor Compagna ce ne fa lezione - esso serviva, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione, a collegare il Parlamento con il Governo. Il Governo, nominato dal Presidente della Repubblica, doveva,

Da ultimo, ad esempio, il fatto che si sia traviata la sostanza dell'articolo 94 della

ha fatto votare il popolo, proprio in funzione della materialità della Costituzione, per la quale veniva assunta l'esistenza di un'investitura diretta del Presidente del Consiglio. Ciò che succede oggi, con una continua una continua apposizione della questione di fiducia, costituisce ancora di più una richiamata novazione materiale della Costituzione, perché la continua apposizione della questione di fiducia richiama quei Governi presidenziali,

Oggi invece il Governo ci ha abituati all'apposizione della questione di fiducia, che è una novazione materiale alla quale il Governo fa riferimento. Allora non si può dire che il Governo è eletto dal Parlamento e poi contemporaneamente richiamare delle prerogative che ovunque in dottrina sono attribuite ai Governi presidenziali, che ricevono un'investitura popolare. Con la continua apposizione della questione di fiducia il Governo determina una bipolarità di conduzione nel rapporto tra Governo e Parlamento

Se non vogliamo citare De Curtis e vogliamo citare qualcosa di più aulico, diciamo che quello che succede nel votare oggi una mozione di sfiducia *ex* articolo 94, differentemente da quello che succede quando il Governo pone una questione di fiducia,

In questo caso, invece, non condividiamo la base sulla quale è posta la mozione di sfiducia, ma finiamo a prescindere per votare contro il Governo.

Se la posizione di autonomia del Gruppo verrà dichiarata al momento del passaggio sotto il banco della Presidenza, possiamo tranquillamente dire che il Governo non ha di che preoccuparsi dal voto di quest'Assemblea. Quello che sta avvenendo, come un po' arrogantemente ha detto il Governo, non è altro che una mera affermazione di principio: il Parlamento prende occasione, non potendolo altrimenti fare su provvedimenti su cui il Governo pone la questione di fiducia, di discutere della politica del Governo, ma finisce per dare a questo voto un significato che è una mera affermazione di principio.

quando, forse presto, esprimerà la vera ed unica sentenza passata in giudicato sull'operato del Governo. Un operato che noi non giudichiamo affatto tale da poter avere la nostra fiducia.

Ho sentito, nelle parole di Matteo Renzi, riecheggiare concetti cari a Mino Martinazzoli e a Benigno Zaccagnini

anche il successivo dibattito che, per prassi parlamentare in sede di dichiarazioni di voto, deve necessariamente svolgersi. Mi chiedo perché noi siamo qui. Di cosa stiamo discutendo? Di una serie di mozioni di sfiducia che hanno preso l'abbrivio da un fatto di cronaca, ovverosia dalla pubblicazione di intercettazioni che, in un primo momento, sembravano coinvolgere il ministro Guidi ma che, successivamente, per intervento chiarificatore della magistratura, hanno inequivocabilmente dimostrato che il ministro Guidi era parte lesa e non aveva partecipato a quel traffico di influenza. Anche questo è un reato che ci siamo inventati in queste Aule, per consentire a certa magistratura politicizzata di mettere le manette allo sventurato politico di turno. E di questo non possiamo che pubblicamente dolerci. Mancano quindi i presupposti che hanno dato fiato alla variegata orchestra delle opposizioni.

la morale risiede nella legge. Lo Stato è un ente collettivo e non può orientare le proprie scelte se non attraverso le leggi che promulga e al cui imperio devono soggiacere tutti i cittadini. Quella è l'etica pubblica. In questa Nazione, dove la politica si è rarefatta e segue l'andazzo dello scandalismo di piazza, dove i parlamentari debbono subire questa involuzione e diventare semplici portavoce dei cittadini (a quanto pare), il Parlamento si anima sulla scorta, non di problematiche attinenti al Governo e alla vita della Nazione, ma sotto la spinta "gossipara" di una stampa che, per molti versi, non è più interessata all'informazione ma allo scandalismo, a fare il catenaccio cubitale, per infarcire poi l'articolo di una serie di illazioni, di congetture, di veline sottratte a dei pubblici ministeri un po' sbadati, ma che continuano a non pagare il fio della propria sbadatagine. Pertanto, si alimenta ancora di più la macchina del fango, la macchina pretestuosa e capziosa di coloro che pensano di poter seguire la scorciatoia di eliminare il governante di turno, l'avversario politico di turno, sotto il peso delle nefandezze che il circuito mediatico giudiziario mette in piazza. piazza. La morale dei singoli, che è quella serie di comportamenti e convincimenti che appartengono ai singoli individui, viene scambiata e contrabbandata come etica pubblica.

Di cosa dobbiamo parlare? Dei mal di pancia di chi si vede oggi costretto a inseguire il *gossip* di coloro che scambiano la politica con l'esercizio di raccogliere cenci sporchi nella pattumiera della maldicenza? Su quale base noi dovremmo assentire a mozioni di sfiducia che non hanno né motivazione etica, né motivazione politica?

ci narra. La mitologia greca ci racconta che Zeus consegna ai suoi fratelli Prometeo

i poteri che consentono agli individui che stanno sulla terra di poter sopravvivere al caos. Epimeteo fa tale distribuzione agli animali:

vede prima), per evitare che le belve che sono state dotate di poteri possano divorare gli uomini, ruba il fuoco, perché attraverso il fuoco

sono divisi, non sono organizzati e quindi protetti dalla malvagità delle belve e dalle insidie della natura. Pertanto Prometeo ruba la *politiké tèchne,* cioè l'arte della politica, ovvero quella serie di regole che consentono all'uomo di vivere in società, di costituire una comunità, di costruire lo Stato.

caleidoscopica, multiforme che da una società di individui può venire per garantire la civile convivenza.

Karl Popper ci ammoniva dicendo che la democrazia non consiste nel sapere chi deve comandare (questo lo decidono gli elettori); sosteneva che non è importante sapere se deve comandare Calderoli o Renzi. L'importante è sapere che la democrazia funziona perché Calderoli o Renzi possono essere assoggettati alla più incessante critica, perché se non c'è la critica c'è il monopolio delle idee, c'è il pensiero unico, c'è la dittatura. Questo principio di critica deve tuttavia fondarsi sulla *tèchne* politica, cioè sul principio si muovono le critiche all'interno di regole consustanziali alla politica, non di evanescenti ed estemporanee iniziative che non servono che a buttare fango su chi deve governare. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, chiedendo scusa forse del pistolotto, che il senatore Centinaio certamente non avrà gradito; spero almeno che lo abbia compreso. Oggi noi abbiamo ascoltato un Presidente del Consiglio che ha avuto il coraggio e gli attributi per distinguere tra giustizia e giustizialismo; ha avuto il coraggio di dire in quest'Aula quello che molti imbecilli (da *imbaculus*, uomo senza bastone, senza carattere) ripetono nei corridoi; soprattutto però ha dimostrato di non essere un idiota. Idiota deriva dal greco e significa uomo isolato, uomo avulso dalla realtà, dal contesto; egli non è stato un idiota: si è calato dentro i problemi, ha dato delle risposte, lo ha fatto con coraggio e non credo che qua dentro di idioti ce ne siano più di un centinaio. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, oggi siamo di fronte all'ennesimo ricorso all'istituto della mozione di sfiducia, questa volta nei confronti del Governo nella sua interezza. Ebbene, non si può non notare la totale assenza di ogni reale contenuto e l'assenza di uno schieramento coeso che possa sostenerli. La dice lunga che le opposizioni non siano nemmeno riuscite a mettersi d'accordo su un testo comune. L'unico punto di accordo delle opposizioni è, a quanto pare, la disperata ricerca di una maggioranza favorevole alle dimissioni del Governo. Si tratta, quindi, di una finalità esclusivamente distruttiva, senza che le opposizioni siano in grado di offrire una valida alternativa.

che ogni forza parlamentare ha nei confronti del Governo. Come Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE non abbiamo alcun motivo per contraddire il patto di maggioranza con il Governo Renzi. È un Governo che, a nostro giudizio, ha operato bene dimostrando sensibilità anche nei confronti delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali. Dopo una lunga fase di stallo durante i precedenti Governi di centrodestra e del Governo Monti, con questo Esecutivo siamo finalmente riusciti a risolvere molte questioni importanti per le nostre autonomie. notevolmente il contenzioso tra lo Stato e le Regioni, anche ordinarie, davanti alla Corte costituzionale che, sotto i precedenti Governi, aveva raggiunto livelli molto preoccupanti. Condividiamo anche le posizioni che il Governo ha assunto per quel che riguarda le politiche di controllo dei flussi migratori. Il presidente Renzi ha fatto bene a fare proposte concrete per una politica europea di immigrazione comune. Si oppone giustamente ad un'Europa delle barriere e degli egoismi nazionali. Ha annunciato di non voler tollerare la violazione delle regole di Schengen che potrebbero derivare, in particolare, dall'eventuale chiusura del confine del Brennero. Questo Governo sta attuando quello che ha promesso ai cittadini al momento della sua nascita, ossia un ambizioso programma di profonde riforme economiche ed istituzionali. In meno di due anni questo Governo è riuscito a fare tanto, in primo luogo ad approvare riforme di assoluto rilievo, come viene riconosciuto in Europa e dai maggiori organi ed istituzioni internazionali. Chi di noi avrebbe pensato nel 2014 che Renzi e questa fragile maggioranza - come all'inizio si è presentata - sarebbero in grado di dare al Paese una nuova legge elettorale, di modernizzare il mercato del lavoro, di ridurre in modo significativo le tasse sul lavoro e di approvare una riforma costituzionale e, quindi, di fare le riforme attese da decenni? Vale la pena ricordare che solo per questi indubbi successi sia stato possibile beneficiare delle clausole di flessibilità che hanno consentito all'Italia, con l'aiuto della mirata Voi, cari colleghi dell'opposizione, volete mandare a casa un *Premier* con questi risultati senza aver peraltro una credibile alternativa?

che la classe politica italiana prosegua con le riforme e con il lavoro costruttivo per il progresso e il benessere del Paese. Credo che tutti sappiano che non esiste una maggioranza parlamentare contro questo Governo, per cui anche questa mozione di sfiducia - anziché mettere a rischio l'Esecutivo - lo rafforzerà. Oggi ci sarà quindi il secondo *flop* delle opposizioni nel giro di soli due giorni; anche questo è quasi un Come se non bastasse l'insuccesso di domenica scorsa, dove avete cercato di snaturare e strumentalizzare lo strumento *referendum* popolare per fini che avevano nulla a che fare con il quesito sottoposto ai cittadini. I cittadini sanno, invece, ben distinguere tra chi strumentalizza e urla e chi è invece disposto ad assumersi la responsabilità di lavorare per il bene del Paese. Noi non condividiamo questa tendenza irresponsabile di voler sfiduciare il Governo ogni settimana. Lasciamo lavorare Renzi e la sua squadra, perché c'è ancora tanto da fare. Poi - nel 2018 - saranno i cittadini a giudicare. Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE voterà contro le mozioni di sfiducia presentate.

Grazie a tutte basata su energie pulite e rinnovabili, queste sì in grado di creare molti posti di lavoro. Per questo, anche se il *quorum* non è stato raggiunto, quel voto non è stato affatto inutile e non potrete non tenerne conto. Si è votato, però, anche contro l'arroganza di un Capo di Governo che, caso più unico che raro, incita all'astensione. Per questo si è accusato i referendari di strumentalizzazione politica. Ma è lei, Presidente del Consiglio, che ha fatto questa operazione, mettendosi al centro dello scontro con l'invito a disertare le urne, per trasformare in modo truffaldino l'astensione, ormai attestata su livelli patologici per la nostra democrazia, in consenso, scommettendo così di fatto sull'erosione della partecipazione e quindi della democrazia. Il 70-30 di cui lei ha parlato indica chiaramente questo. Rivendicando quel risultato come un suo successo lei si pone, in una torsione pericolosa, come una specie di capo della maggioranza silenziosa e non votante. Come scrive lucidamente oggi Diamanti nella sua analisi del voto, è inquietante che lei, Renzi, veda nell'astensione una risorsa, una fonte di consenso politico e personale. Ma questa, come abbiamo ripetuto più volte, è la strada su cui lei si è incamminato da tempo, tentando di fare del *referendum* costituzionale un plebiscito e in realtà trasformando tutto in un *referendum* su di sé, tranne le prossime amministrative, guarda caso. Ma, d'altronde, è la trasformazione del nostro sistema democratico e della forma di Governo che lei sta perseguendo da tempo e che è la sostanza della sua revisione costituzionale: il Governo del *Premier*.

perché molti elettori avrebbero fatto facilmente due più due: si sarebbero accorti delle affinità tra un emendamento che regala a Total e Shell la possibilità di devastare ulteriormente una città già piegata dall'ILVA come Taranto - senza alcun vantaggio, sia ben chiaro, per il nostro Paese e una norma che permette alle stesse compagnie di risparmiare un miliardo di euro non smantellando gli impianti e le piattaforme che, ormai si sa, almeno per la metà sono inattive. E, come se non bastasse, tenendosi, Grazie a tutte chi conosce le «meraviglie» dell'estrazione petrolifera, vorrebbe volentieri e con forza evitarle. Il *quorum* non si è raggiunto, ma non credo lei abbia molte ragioni per gioire, e prima di tutto perché la legge sulle concessioni senza termine contrasta con il diritto comunitario, come ho segnalato nella denuncia che ho sporto presso la Commissione europea, e l'Italia sarà certamente soggetta a procedura di infrazione. Soprattutto, lei non ha alcun motivo di soddisfazione perché, nonostante i 300 milioni buttati buttati per evitare che il *referendum* fosse accorpato alle amministrative - voi li avete buttati - nonostante il ricatto bugiardo sui posti di lavoro e nonostante aver voluto bypassare anche questo dibattito, 13,5 milioni di italiani si sono recati alle urne per dire sì a una politica energetica opposta a quella che lei fa in concreto e che è ben diversa da quella che va sbandierando pubblicamente, possibilmente all'estero. Esaltare le energie alternative per farsi belli in TV o nelle battute che ha fatto oggi e, allo stesso tempo, tagliare i fondi per quelle medesime energie rinnovabili è un'ennesima truffa. Vi ricordo cosa avete fatto con il decreto cosiddetto spalma incentivi. In queste settimane l'inchiesta che ha già costretto alle dimissioni l'ex ministro Guidi non si è affatto ridimensionata. Al contrario, appare oggi ancora più grave di quanto non fosse poche settimane fa. È indagato il vicepresidente di Confindustria, il sottosegretario De Filippo; è stato confermato il sequestro dell'impianto ENI di Viggiano. Dopo il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio De Giorgi, è finito sotto inchiesta anche un altro ufficiale della Marina, il contrammiraglio Berutti Bergotto. Spetta certamente alla magistratura accertare le responsabilità penali e noi, al contrario di lei, signor Presidente del Consiglio, non scopriamo il garantismo oggi, e non lo abbiamo mai utilizzato a seconda se eravamo in maggioranza o all'opposizione. In realtà, quello che oggi vogliamo sottolineare - e che politicamente è chiaro - è che intorno all'infrastrutture di Taranto e di Augusta si agitava un gruppo di interesse forte, di relazioni potenti all'interno del Governo; un gruppo, anzi - per adoperare il termine usato dall'*ex* ministro Guidi - una cricca di furbetti

non spetta a noi decidere sulle eventuali responsabilità penali. Questo è compito della magistratura. Spetta però al Parlamento giudicare quel che da questa vicenda - e non solo da questa - è emerso e sta emergendo sotto il profilo della responsabilità politica. Da questo punto di vista, politico e non penale, un giudizio definitivo è possibile già oggi, anzi è doveroso. Se sommiamo questa vicenda a quella precedente del salvataggio delle banche più o meno di famiglia e ai criteri con i quali vengono fatte le nomine, ci troviamo di fronte a un quadro nel quale i conflitti di interesse proliferano. Vengono sfornate leggi che toccano direttamente interessi di parenti stretti; le nomine vengono decise con il criterio della prossimità con il Presidente del Consiglio o con la sua cerchia. Non è facile trovare altrettanti esempi nella nostra storia. Non è certo una coincidenza se, con un Governo in cui i conflitti di interessi sono così numerosi e marcati, la legge che dovrebbe risolvere quei conflitti, approvata dalla Camera e ora all'esame della 1a Commissione qui al Senato, risulta per l'ennesima volta annacquata, inadeguata a fronteggiare un problema che ormai da decenni grava sulla politica italiana. Ci sono i parenti e gli amici, ma ci sono anche, e a maggior ragione, gli interessi dei gruppi di potere, che conviene tenersi buoni. Dall'inchiesta in corso emerge con chiarezza l'attività febbrile e incessante delle *lobby*, impegnate nel condizionare le scelte del Governo a vantaggio dei loro interessi a scapito del bene pubblico e dell'interesse dei cittadini. Questa attività si è esercitata con ogni mezzo: scambio di favori, pressioni continue per ottenere la nomina di amici affidabili e disponibili nei posti chiave, vincoli privati fatti valere a peso d'oro. È

Tutto ciò sarebbe di per sé estremamente inquietante. Sappiamo tutti che, quando il lobbismo arriva a questo livello estremo di intensità, è segno che sa di poter raggiungere i propri obiettivi. Ma il peggio è che allo sforzo delle *lobby* corrisponde una permeabilità estrema del Governo. L'elemento davvero scandaloso

legge di stabilità al Senato e viene così approvato col voto di fiducia. L'elemento inquietante non è che un faccendiere si faccia in quattro per ottenere la nomina di Alberto Cozzo come commissario del porto di Augusta, ma che il ministro Delrio lo nomini davvero. È del tutto evidente che siamo qui di fronte a un atteggiamento complessivo dell'intero Governo, e in particolare di Palazzo Chigi, dove è stato messo a punto l'emendamento che Total e Shell esigevano. Per questo le dimissioni, pur doverose, del ministro Guidi non bastano affatto per chiudere la vicenda. È l'intero Governo, primo fra tutti lei, Presidente del Consiglio, che dovrebbe rassegnare le dimissioni;

la sudditanza ai voleri delle *lobby*, il trasformismo, come quello su cui si basa la sua maggioranza parlamentare, sono antichi come la peggior Grazie a tutte Ma dovrebbe sapere che si possono ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo, ma non si riesce mai, alla fine, a ingannare un popolo. Lei lo ha ingannato abbastanza. Per questo, Presidente del Consiglio, noi voteremo a favore della mozione di sfiducia al suo Governo. Presidente, il nostro Gruppo voterà contro le mozioni di sfiducia presentate nei confronti dell'Esecutivo e vorrei partire dagli eventi che hanno dato luogo alla loro presentazione, analizzando analizzando i contorni politici e le eventuali anomalie che potranno esserci di valido ausilio per il dopo. Le dimissioni del ministro Guidi hanno sicuramente reso più sereno il clima politico che si era determinato attorno all'inchiesta della procura di Potenza, ciò ci consente oggi di riflettere meglio su alcuni aspetti che possono costituire spunto per interventi legislativi in materie delicate come la regolamentazione delle *lobby*, il conflitto d'interessi, le intercettazioni e la durata dei processi. In Italia manca una disciplina legislativa che regolamenti l'esercizio dell'attività lobbistica, vista nella sua corretta accezione di dialogo e confronto tra le rivendicazioni e le esigenze di corpi sociali e produttivi - da un lato - e potere legislativo ed esecutivo, dall'altro. Tutto ciò porta a contatti diretti di rappresentanti di categoria con il mondo della politica e del Governo: nessuna barriera, nessun filtro, nessuna selezione. Occorrerà, allora, provare a individuare meccanismi che assicurino un confronto tra l'Esecutivo ed il privato attraverso regole di rigida trasparenza, pubblicità e tipicità delle procedure da adottare. Dico questo non perché mi manifesti contrario al dialogo tra Stato e cittadino, ma perché penso che dobbiamo, per il futuro, attraverso un'eventuale disciplina delle attività di *lobby*, sgombrare il campo da qualunque sospetto di presunte ingerenze del privato sul pubblico. Il tema di questa disciplina ci porta all'esigenza di una rivisitazione della normativa sul conflitto d'interessi, quando, essendo portatori di interessi specifici derivanti dalla propria attività, si è chiamati a ricoprire cariche di Governo o parlamentari. Ma il problema, signor Presidente, si accentua ancora di più quando rappresentanti nazionali di categorie imprenditoriali estese su tutto il territorio ricoprono ruoli parlamentari.

abbiamo assistito per l'ennesima volta alla pubblicazione di intercettazioni telefoniche che, prive di rilevanza penale, hanno coinvolto soggetti estranei ai fatti delittuosi, facendoli apparire come soggetti concorrenti nel reato. Non è bello vedere pubblicato il proprio nome in un quotidiano solo perché esso risulta trascritto o citato incidentalmente nell'inchiesta e assistere passivamente, attraverso quella pubblicazione, a un processo di condanna mediatica nei suoi confronti senza alcuna colpa o responsabilità. E non è bello, all'indomani di questi eventi che si ripetono con sistematica periodicità, assistere al coro degli indignati per la palese e grave violazione della *privacy* e, a volte, alla condanna mediatica che ne deriva; cori accompagnati dagli intenti di indifferibili modifiche legislative che evitino questi inaccettabili scenari, per poi veder spegnere nel tempo queste indignazioni che si richiudono nei cassetti. Noi siamo pronti a condividere immediatamente una legge che, lungi dal limitare l'utilizzo delle intercettazioni ai fini investigativi, ne limiti forme di pubblicità inopportune, evitando il deposito negli atti di indagine di quelle del tutto prive di rilevanza penale.

perché nessuno può escludere che altre procure non ritengano di adottare questi codici di comportamento. E non si dica, per favore, che si vuol imporre una legge bavaglio, perché l'obiettivo dovrà essere quello di una legge di civiltà a tutela del cittadino e della giustizia. Ella, signor Presidente del Consiglio, ha auspicato tempi più veloci per le sentenze. Non posso che condividere e sottoscrivere pienamente il richiamo del Presidente del Consiglio, perché in ciò ritrovo quel principio della presunzione di innocenza previsto dalla nostra Costituzione e troppo spesso oscurato da campagne mediatiche o movimenti di opinione pubblica che portano a sentenze di condanna preventive, ingiuste e inaccettabili. Il signor Presidente del Consiglio ha invocato la celerità nei processi e le relative sentenze proprio per evitare questi scenari. Ma attenzione, perché questo tema e questo obiettivo - secondo me - troverebbero un ostacolo insormontabile con l'eventuale scelta di prolungare i termini di prescrizione del reato. La conseguenza di tale scelta sarebbe, infatti, la inevitabile dilatazione dei tempi di durata dei processi, e noi siamo contrari ad avallare la figura dell'"imputato a vita". Sono convinto che, se vogliamo sentenze celeri, dobbiamo intervenire attraverso l'introduzione di nuove regole rigide che fissino tempi certi e inderogabili per tutte le fasi processuali e, in particolar modo, per quelle relative alla durata delle indagini, in quanto proprio la lunghezza, a volte eccessiva, di quest'ultima fase, dove l'attività difensiva è inibita e quindi non può essere considerata causa di effetti dilatori, porta poi i processi vicini alla prescrizione già nella prima o nella seconda fase dibattimentale. II principio della prescrizione, signor Presidente, obbedisce a due esigenze: la prima è quella di garantire al cittadino tempi certi per la durata di indagini e processi a suo carico, evitandogli quindi il calvario di una qualità della vita spesso offuscata o appesantita dai dubbi o preoccupazioni di un procedimento a suo carico quando questi poi in effetti si riveli innocente. La seconda esigenza è quella di evitare all'imputato di doversi difendere da fatti storicamente troppo lontani rispetto all'avvenuta contestazione e per i quali, quindi, possa configurarsi difficile da parte sua il rinvenimento di prove a discarico. E in questo solco io credo si ponga mirabilmente l'articolo 111 della Costituzione nella nuova formulazione della legge costituzionale del 1999, della quale è stato ispiratore il nostro collega Marcello Pera e votata da questo Parlamento, signor Presidente, quasi all'unanimità. Parliamo della «ragionevole durata del processo», principio scolpito indelebilmente in Costituzione, che verrebbe violato da una norma che, dilatando i termini di prescrizione, determinerebbe innegabilmente la dilatazione dei tempi processuali. Sul testo della prescrizione esitato dalla Camera il mio Gruppo non ha votato contro ma si è astenuto, a seguito delle assicurazioni del ministro Orlando di modifiche al Senato. E noi, in assenza delle modifiche promesse, saremo coerenti in assenza delle modifiche promesse, saremo coerenti con il pensiero dei nostri colleghi deputati, e respingeremo al mittente le eventuali critiche di chi ci dovesse contestare di volere l'impunità dei colpevoli. La nostra storia politica ci ha visti protagonisti, in passato, di forti iniziative legislative contro ogni forma di illegalità. Cito tra tutte, quelle contro la criminalità organizzata. Lo abbiamo fatto nel 2002, con la stabilizzazione dell'articolo 41-*bis* da me proposta, e con l'approvazione, nel 2013, della norma sul sequestro per equivalente, da me suggerita e caldeggiata durante la trattazione del pacchetto sicurezza in Senato, e condivisa e sostenuta dal ministro della giustizia dell'epoca, Angelino Alfano, il quale, tra l'altro, in quell'epoca ha anche inasprito il regime del 41-*bis*. E, nell'approvare queste norme, non abbiamo fatto proclami, ma abbiamo valorizzato il fatto della loro unanime condivisione parlamentare, perché si commette un grave errore, colleghi, quando le forze politiche si dividono strumentalmente nella lotta alla mafia. Le si farebbe un favore. La mafia si combatte con i fatti, con le leggi e le coraggiose indagini della magistratura, e poco invece con quegli atteggiamenti di una antimafia fatta di proclami, interviste e carriere costruite su immagini di forti tutori della legalità, che proprio in questi ultimi periodi - mi spiace doverlo dire - si stanno a volte rivelando dense di zone d'ombra significative e inquietanti. Signor Presidente, la nostra è un'alleanza complessa, ma responsabile, perché è frutto di un'intesa di Governo tra due forze politiche con storie diverse, con corpi elettorali di provenienza diversa, con collocazioni europee diverse, con valori a volte di difficile conciliabilità. Un principio, comunque, ci accomuna: il rigetto di ogni forma di estremismo o populismo. Ciò non ci ha, però, impedito di realizzare importanti obiettivi del nostro programma: il *jobs act*, il patto per la salute, il "no" all'IRAP nel costo del lavoro, le zero tasse nel triennio per i neo assunti, l'ecobonus, padroni in casa propria, la legge contro la violenza di genere, lo sblocco dei tetti stipendiali per le nostre donne uomini in divisa, la legge contro la violenza negli stadi. Ci batteremo per più incisive misure di sostegno alla famiglia e al Mezzogiorno; per una politica economica aggressiva dell'enorme debito pubblico, che non accenna a diminuire, e una conseguente riduzione della pressione fiscale; per un aumento degli investimenti pubblici e la semplificazione di tutte le relative procedure. Lo faremo dialogando responsabilmente all'interno della maggioranza, nell'auspicio che al Senato vengano assegnati giusti tempi di dibattito, recentemente sottrattigli in occasione di recenti decreti-legge di riforme strategiche. Mi accingo a concludere, signora Presidente. però intransigenti su alcuni principi, quali il garantismo, la meritocrazia, la trasparenza nelle scelte di figure esponenziali, il valore della vita e della famiglia prevista in Costituzione, la genitorialità eterosessuale. Alcune settimane or sono si è evitata una forte lacerazione nella maggioranza a proposito della norma sulla *stepchild*. Noi non siamo arretrati di un millimetro, così come mai arretreremo tutte le volte in cui si cercherà di mettere in discussione i principi irrinunciabili della nostra identità. un'identità che ci vede anche tutori del principio dell'accoglienza di chi fugge dalla guerra e dai genocidi, ma strenui difensori della legalità e della sicurezza dei nostri confini e del nostro Paese, che oggi è chiamato a contrastare un nuovo e terribile nemico invisibile qual è il terrorismo, che il nostro Governo quotidianamente combatte in silenzio e con grande professionalità. Tale compito è svolto anche e soprattutto grazie all'encomiabile lavoro quotidiano di donne e uomini delle Forze dell'ordine che assicurano, a rischio della loro vita, sicurezza alle nostre famiglie e ai luoghi. A loro, sentitamente, va il nostro ringraziamento. Grazie di cuore! solo un appunto, prima di iniziare il mio discorso. Il presidente Renzi ha dato del "maleducato" ai senatori. Vedo che qui manca tutto il Governo, compreso il presidente Renzi,

tutte le "non riforme" che ha fatto, compresi i risultati non reali sulla nuova occupazione, in quanto il numero di cui ha parlato - i 950.000 contratti

Grazie a tutte

quest'Aula del Parlamento deve fare i conti con lo scandalo enorme che da settimane ha travolto il Governo. La Trivellopoli di oggi è paragonabile alla Tangentopoli del 1992, quella Tangentopoli che travolse Governo e istituzioni italiane esattamente come oggi questa marea nera, nera come il petrolio, sta sommergendo il vostro Governo, il PD e i suoi illustri esponenti. Da Tangentopoli e dall'inchiesta di Mani pulite sono passati più di vent'anni, ma oggi come allora dobbiamo prendere atto che le istituzioni italiane e questo Governo, in particolare, non sono stati in grado di rendersi impermeabili alle infiltrazioni della corruzione e del malaffare e non hanno voluto risolvere i propri conflitti di interesse e resistere alla tentazione di piegare la politica a strumento di potere e di indebito arricchimento personale. E, quando il malaffare penetra istituzioni e Governo, è perché Governo e istituzioni sono permeabili alle infiltrazioni e dunque complici. Oggi, esattamente come in quei bui anni Novanta, la cosa pubblica è ancora cosa loro. Per raccontare Trivellopoli è utile partire dai reati che la procura di Potenza e l'antimafia contestano agli indagati.

concussione, induzione indebita, truffa aggravata per erogazioni pubbliche, traffico illecito di rifiuti e miscelazione di rifiuti speciali, abuso d'ufficio.

l'ex ministro Guidi, le cui dimissioni sono state un atto dovuto, che però non salva la faccia all'intero Esecutivo; il ministro per le riforme Boschi; il ministro delle infrastrutture Delrio; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti; il sottosegretario alle infrastrutture Vicari; il presidente della Regione Basilicata PD); il capo segreteria della senatrice Finocchiaro, Paolo Quinto. Poi ci sono gli indagati: il sottosegretario alla salute De Filippo; il consigliere regionale

Questa inchiesta ci racconta di un sistema di potere marcio e ipocrita, con istituzioni manovrate da una cricca, un clan, un quartierino, un'associazione a delinquere che muove Ministri e Ministeri come pedine su una scacchiera, Grazie a tutte svela a tutti gli italiani come avete operato e perché oggi le vostre mani sono sporche e grondano petrolio! *(Commenti dal Gruppo PD)*. In pieno conflitto di interessi, avete lavorato per favorire multinazionali come la francese Total, a danno della salute dei cittadini della Basilicata e dell'ambiente. Sblocca Italia e legge di stabilità sono servite come cavalli di Troia per inserire di nascosto norme spinte dalla cricca che faceva capo al compagno dell'*ex* ministro Guidi, norme che sbloccavano l'impianto di Tempa Rossa e in un colpo solo tagliavano le autorizzazioni necessarie per portare il petrolio estratto in Basilicata fino a Taranto, dando l'ultima parola al Governo e disattendendo la volontà di Regioni, Comuni e cittadini. Chi ci guadagna in questa operazione? Gli italiani? I cittadini lucani che si ammalano di tumore? I territori inquinati dagli sversamenti dei pozzi di petrolio? Certamente no! Mentre il Paese fa fatica a ripartire e a risollevarsi, avete permesso alla cricca del petrolio

tu mi fai fare l'emendamento sblocca petrolio e io ti do il subappalto da 2,5 milioni di euro; tu mi nomini il commissario dell'Autorità portuale

speculato sulla salute dei cittadini, sulla difesa e sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente e del nostro territorio e, cosi facendo, avete perso ogni brandello di dignità e credibilità. Colto con le mani nel petrolio prima dal Movimento 5 Stelle, poi dalla procura della Repubblica, il presidente Renzi ha rivendicato il famoso emendamento Tempa Rossa, come se mettere i piedi in testa alle Regioni e ai cittadini che in quei territori ci vivono e sbloccare un'opera privata da cui l'Italia non ricaverà un fico secco fossero un vanto o una medaglia da appuntarsi Ma questa medaglia - e ve lo dico col cuore in questa Aula - signori, viene pagata a caro prezzo, con le vite della gente che vive in Basilicata e muore a causa dell'inquinamento. Guardatele! Andateci!

tutti i suoi ministri, *in primis* il ministro Boschi che ha permesso che l'emendamento marchetta sponsorizzato dalla Guidi entrasse nella legge di stabilità. Il Movimento 5 Stelle è orgoglioso di aver denunciato il marcio che oggi è sotto gli occhi di tutti. Siamo andati in Basilicata, siamo stati ad Augusta. Ieri ho trascorso un'ora a con don Palmiro Prisutto, quel parroco coraggioso che ogni 28 del mese ad Augusta denuncia ed elenca i morti di cancro e di tumore. Trivellopoli è solo l'inizio, così come all'epoca l'arresto è solo l'inizio, così come all'epoca l'arresto di Mario Chiesa fu soltanto l'antipasto della valanga che poi sarebbe arrivata con Tangentopoli. Trivellopoli è la punta di un *iceberg*. Gli italiani devono sapere con chiarezza che la mozione di sfiducia sarà bocciata da quest'Aula per un motivo molto semplice: il Gruppo del senatore Verdini - gli amici di AL-A, come li chiama il presidente Renzi - che è proprio quello che ieri è stato rinviato a giudizio per la sesta volta in due anni

CATALFO *(M5S)*. Corruzione e malaffare, in quest'Aula, si nutrono, si salvano e si autoassolvono: uno spettacolo indegno per un Paese civile! Delinquenti penali supportano (e salvano) delinquenti politici. Siete gente senza pudore

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il marchese del Grillo si è ritirato nel suo palazzo e noi - la citazione è nota - che poco siamo, siamo qui.

tutte le truppe del Governo, ed è rimasto solo qualcuno che deve votare; giustamente qualcuno è tornato perché, essendo senatore, deve votare, e quindi sono anche fortunato, ma è una circostanza e non un gesto di considerazione verso le opposizioni.

perché il Governo, che si era presentato come quello dei rottamatori, degli innovatori, dei candidi nuovi soggetti della politica, poi in realtà, dopo un tempo non lunghissimo, si è trovato invischiato nei classici argomenti un po' untuosi,

mesi a doversi giustificare per quello che è successo nelle banche popolari e in Basilicata, dove a noi è sembrato che il petrolio, invece di trovarlo gli italiani, lo abbia trovato il Partito Democratico. Noi non veniamo meno alla nostra posizione garantista e, quindi, certamente attendiamo l'esito delle vicende giudiziarie. Noi abbiamo sottoscritto una mozione di sfiducia che potremmo essere portati a definire una sfiducia alla carriera e, quindi, al complesso degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle condotte del Governo Renzi. Per quanto riguarda il tema del garantismo, dobbiamo dire una cosa, e me lo consentirà il presidente Napolitano con rispetto, ma anche con la franchezza del nostro argomentare. è matura la condizione per fare una legge sulle intercettazioni. Presidente Napolitano, era matura anche qualche anno fa, quando non abbiamo potuto fare quella legge.

sa, è una regola fondamentale.

presidente Renzi, non c'è solo il senatore Margiotta che ha subito in silenzio processi ingiusti; è capitato a tanti di noi di subire - come abbiamo ricordato in quest'Aula - accuse che non avevano fondamento e le abbiamo affrontate con spirito istituzionale. tuttavia, contestiamo anche il sottobosco di affarismo. Penso che il ministro Guidi, per molti versi, sia stata una vittima e si è anche dimessa e, quindi, si è assunta delle responsabilità per sé e per altri. Ma tutto il sottobosco di Gemelli, non Gemelli, di rappresentanti che dovevano stare al Ministero, anche senza la stanza purché stessero lì, ha rappresentato uno spaccato che un Governo come questo, di rottamatori e innovatori, non doveva avere, perché è qualcosa di molto antico, di molto classico, di molto desueto, essendoci sempre stati questi tipi di personaggi che vanno messi al bando. Vedremo quali saranno colpevoli quali saranno innocenti. Non abbiamo nemmeno partecipato, come Forza Italia, a un coro di denigrazione delle Forze armate, perché a questo non ci siamo mai prestati e non ci presteremo. Semmai, abbiamo da recriminare se i giusti soldi destinati alla legge navale servono a usare le navi per le operazioni che trasportano i clandestini e non per la sicurezza del Paese. Abbiamo semmai da ridire sull'impiego che il Governo impone alla nostra Marina.

perché Renzi - risponda al quesito il candidato - ha chiesto per il 2015 all'Unione europea che si riconoscesse all'Italia uno sforamento di 3 miliardi di euro dai conti pubblici per le spese in più fatte per l'immigrazione? *(Applausi dal Gruppo

un controllo benché ci sia un nuovo Governo che stenta ancora a camminare, ma gli sbarchi sono aumentati e sono migliaia al giorno. Ci vorrebbe il contatore come quello di Telethon quando si raccolgono i soldi per beneficenza, per aggiornare di minuto in minuto il numero degli sbarchi. E anche la missione - lo sa il ministro Pinotti, visto che è argomento di nostra contestazione - EUNAVFOR Med a cui partecipa la nostra Marina doveva servire a combattere gli scafisti. Ma, siccome il Governo libico non è ancora in grado di controllare le coste e le acque territoriali libiche e non ci chiede di intervenire lì, le navi di EUNAVFOR Med partecipano al trasporto di clandestini.

Quindi, il capitolo immigrazione della nostra mozione è uno dei principali motivi di sfiducia. Anche a me da italiano dà fastidio quando l'Austria ci minaccia, ma ricordatevi che qualche mese fa anche la Francia di Hollande, che è un esponente del socialismo europeo, la Francia della rivoluzione francese chiuso il confine a Ventimiglia. Ve la ricordate quella vicenda con i clandestini sugli scogli? Aveva detto che la civilissima Francia, governata dai socialisti, poiché in Italia ne entravano troppi, si era stancata di assistere a questo transito. La strategia italiana qual è? Li porto qua, faccio finta di identificarli, mi giro, se ne vanno e poi i problemi saranno dei francesi, degli austriaci, dei tedeschi e degli svedesi. La Francia si è stufata, così come anche l'Austria. Per carità, sappiamo che, se ci fossero vincoli e chiusure, le nostre merci e i nostri commerci sarebbero minacciati e in pericolo, ma allora dobbiamo porre fine

dopo il *referendum* di ottobre - perché spaventare i cittadini prima? - una manovra economica durissima, severissima, causata da conti che non sono a posto. Anche nelle audizioni, un po' noiose ma importanti e da seguire - suggerisco ai colleghi di leggere domani i resoconti o forse sono Grazie a tutte

La ricordate la riforma Biagi? Era la riforma del mercato del lavoro che portò la disoccupazione ai livelli più bassi della recente storia italiana, intorno all'8 per cento. E Biagi fu ucciso in un clima che non voglio ricordare. Presidente, noi diamo sfiducia a Renzi non solo per le vicende di Potenza, ma per il *caos* della riforma della pubblica amministrazione, per i mancati rimborsi alle imprese che devono aver soldi dallo Stato. Ve le ricordate le scuole da rimettere a posto? I tetti cadono ancora. Ricordate tante altre promesse? L'elenco sarebbe lungo e, per quanto riguarda l'emendamento, oggi Renzi ha detto la verità: «Ma come? Abbiamo fatto anche il subemendamento, non ve ne siete accorti?». Certo, e abbiamo votato contro. Il senatore D'Alì del nostro Gruppo prese la parola in quella notte. Non mi scandalizza che si discuta un emendamento alle 4 del mattino; se si lavora in quelle maratone è normale. Il subemendamento, che ha presentato il relatore di quella legge che è in questa Aula, sapete cosa prevedeva, signori ambientalisti della sinistra? Di trasformare il «concerto» per controllare opere come quelle lucane tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo in un «sentito il Ministero dell'ambiente». Quel subemendamento che avete rivendicato è un ulteriore attentato all'ambiente. Ve la meritate tutta la nostra sfiducia.

trattati da tanti senatori; da alcuni a proposito e da altri a sproposito, da alcuni a tono e da altri invece sovratono. Affronterò solo alcuni aspetti politici e istituzionali che considero molto importanti delle due mozioni. Nei primi tre anni di questa legislatura le opposizioni hanno presentato, tra Camera e Senato, 31 mozioni di sfiducia - quasi una al mese nei primi tre anni della passata legislatura ne sono state presentate sette. In termini di aumento abbiamo una lievitazione del 443 per cento, molto maggiore se parliamo del solo Senato, dove negli ultimi tre anni, le mozioni presentate sono state 22 contro una sola della passata legislatura. I Padri costituenti non volevano certamente questa *routine*. sapete chi è - la mozione di sfiducia era «una procedura speciale ed eccezionale non solo per rendere meno instabili i Governi, ma per evitare discussioni all'infinito». Ruini temeva

Ruini diceva che da questo costume ne sarebbe derivata una ferita alla serietà del Parlamento. Questa ferita oggi è stata inferta largamente a questo Senato. Tra le 31 mozioni di sfiducia di questa legislatura molte sono esempi emblematici di strumentalizzazione politica seriale. Ne ricordo una sola: ad appena quattro mesi dall'insediamento del Governo Letta i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle presentarono una mozione nella quale sostanzialmente chiedevano le dimissioni del Governo Letta per non aver attuato i numerosi punti del loro stesso programma. Rileggendo ora quella mozione possiamo trarne degli spunti molto curiosi. La perla più bella è la richiesta di dimissioni del Governo Letta per non aver abolito l'IMU sulla prima casa.

il Governo Letta lo ha abolito addirittura con decreto-legge, ma anche quella voto volta i senatori del Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Sono due casi che non hanno bisogno di alcuna parola di commento: si commentano da soli. Ora, la degenerazione dell'istituto della mozione di sfiducia, che i Costituenti volevano eccezionale, ha un significato molto chiaro: è un segno inequivocabile delle difficoltà di un'opposizione senza programma, che si è rassegnata alla politica dei 75 milioni di emendamenti da algoritmo, delle pregiudiziali di costituzionalità su tutti - dico della continua richiesta di numero legale, delle uscite in massa dall'Aula, delle contestazioni alla Presidenza dell'Assemblea, delle urla in Aula (che abbiamo sentito anche questa sera, ripetutamente). Nei primi settant'anni di democrazia parlamentare repubblicana le mozioni di sfiducia venivano presentate per fatti molto gravi, quando si pensava che potessero far cadere il Governo o far sciogliere sciogliere le Camere e provocare le elezioni anticipate. Oggi non è più certamente così: nessuna delle forze politiche che ha sottoscritto le due strumentali mozioni che stiamo discutendo vuole l'immediata caduta del Governo, tantomeno le elezioni anticipate, che invece non vogliono (anzi, io credo che temano). Sono iniziative antisistema, con l'obiettivo di ricavarne un titolo sui quotidiani o un passaggio sui telegiornali: solo che il Parlamento non è un *talk* *show* e le mozioni di sfiducia dovrebbero essere una cosa più seria. Ho letto attentamente le mozioni e le ho trovate prive di argomenti che anche solo alla lontana meritino una crisi di Governo. Le mozioni confermano l'impressione che il vero dibattito politico di cui il Parlamento italiano avrebbe oggi bisogno urgente è quello sul modo con il quale le opposizioni fanno politica sia alla Camera, che al Senato. Esaminiamo i fatti. Vi è un'inchiesta giudiziaria ancora in fase istruttoria, che non permette di conoscere gli atti processuali. Non sappiamo se e quali avvisi di garanzia siano stati emessi. Non si ha notizia di rinvii a giudizio. I senatori del Partito Democratico chiedono che l'inchiesta faccia il suo corso con il rigore necessario e senza sconti per nessuno e chiedono soprattutto che il giudizio si celebri. Dico di più. Il Senato sta esaminando la riforma del processo penale, il cui rilievo ai fini di una migliore giustizia e di una più efficace lotta alla corruzione è noto a tutti i senatori. L'indignazione per gli scandali e la richiesta di onestà possono essere sia segni nobili di buona politica sia delle mere intenzioni teoriche. Ma noi siamo senatori della Repubblica e dobbiamo essere capaci di trasformare le indignazioni in buone leggi. Dal contributo di ciascun senatore, dal contributo che noi daremo per portare a casa, bene e rapidamente, la riforma del processo penale si potrà vedere da che parte sta ciascuno di noi. La stampa ha fatto conoscere alcune parti delle intercettazioni telefoniche da cui sono emerse varie forme di disinvoltura verbale e per una di queste conversazioni si è dimessa la ministra Federica Guidi, che peraltro sembra essere parte lesa. In qualsiasi altra democrazia occidentale sarebbero stati immediatamente adottati comportamenti da Stato di diritto: la politica avrebbe dovuto comprendere di dover rispettare la magistratura e attendere le conclusioni dell'inchiesta. Invece, con un riflesso pavloviano, sono immediatamente partite sia la strumentalizzazione politica sia la presentazione delle mozioni di sfiducia. Vedete, di questi tempi la vita politica è molto difficile. Tutti possiamo sbagliare: possono sbagliare la maggioranza e il Governo e può sbagliare l'opposizione. Molti attribuiscono tanta fallibilità alla crisi del sistema politico ed è vero, ma è un'analisi certamente incompleta. la crisi non investe esclusivamente la politica, ma un'intera classe dirigente, e più al fondo intere parti della società. Ed è proprio la profondità di questa crisi planetaria, che è insieme politica, culturale, economica e sociale, a rendere possibili i muri di fil di ferro che stanno distruggendo Schengen, la corsa ai Trump negli Usa, le miopi politiche di rigore e la cecità davanti a fenomeni epocali, come l'immigrazione e il terrorismo. Sono le caratteristiche di questa crisi planetaria che stanno indebolendo le stesse istituzioni e le stesse radici di molte democrazie. Nel Parlamento italiano, però, c'è una differenza molto rilevante: la maggioranza e il Governo possono sbagliare, ma tutte le Cancellerie, tutte le opinioni pubbliche sanno che la nostra intenzione è lavorare per il Paese, per battere la crisi, per assicurare la pace sociale, per difendere l'ideale europeo. Le opposizioni lavorano quotidianamente ed esclusivamente - anche il dibattito di oggi lo ha confermato - per l'interesse della loro parte politica, della loro bottega. E non è una differenza da poco. Fra le democrazie occidentali la nostra è l'unica dove l'azione politica dell'opposizione ha il suo punto di forza non nella contrapposizione di un proprio programma a quello del Governo, ma nell'uso strumentale dei Regolamenti parlamentari con l'obiettivo dichiarato di impedire l'approvazione di qualsiasi provvedimento, persino rischiando di entrare in forte contrapposizione con se stessa, come è successo con l'IMU sulla prima casa e sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Davanti a fenomeni epocali che stanno segnando questo tempo, davanti a flussi migratori biblici, davanti ad un terrorismo internazionale e guerre regionali che fanno parlare di una terza guerra mondiale, davanti ad un'Europa in bilico verso un'inesorabile disgregazione, l'iniziativa politica la trentunesima mozione di sfiducia che già in partenza sanno, dicono, e forse vogliono che venga respinta. Nella giornata nella quale nuovamente piangiamo centinaia di migranti morti nel Mediterraneo, e in cui dovremmo sostenere tutti insieme la bella proposta italiana di sostegno europeo alle Nazioni africane da cui fuggono i migranti, il dibattito sulle mozioni di sfiducia ha qualcosa di veramente surreale. Assistiamo anche a contorsioni politiche che solo poche settimane fa consideravamo impossibili. Il fronte unico delle mozioni vede, oltre alla Lega Nord, ai fittiani e ai 5 Stelle, anche Forza Italia, che ha governato il nostro Paese per tanti anni e che ora si ritrova a fare squadra con quelle forze antisistema che ha sempre detto di detestare. Ma quale prospettiva politica seria può avere una compagnia che in Parlamento va in ordine sparso, salvo mettersi insieme per iniziative sterili e pretestuose? Quale orizzonte politico comune può immaginarsi per Gruppi parlamentari che tra loro si fanno concorrenza e non si tollerano? in democrazia, nessuna maggioranza, nemmeno noi, nemmeno questa maggioranza può rallegrarsi delle difficoltà delle opposizioni. Io non me ne rallegro affatto, e anzi me ne preoccupo perché in democrazia la maggioranza da sola, senza un confronto continuo con un'opposizione vera, non è in grado di garantire un equilibrato sviluppo del Paese. In un sistema politico sano, vivo e vitale, il Parlamento si divide in due parti: maggioranza e opposizione, che, anche se in lotta tra loro, non sono due mondi separati, perché ambedue custodi del buon funzionamento dello Stato, consapevoli che una rottura delle regole danneggerebbe tutti, anche chi l'ha voluta. La stabilità politica è nell'interesse dell'Italia. Dobbiamo quindi augurarci che la legislatura termini alla sua naturale scadenza, e se durerà fino al 2018 - che è un obiettivo né di destra né di sinistra - non potremo certo accontentarci di due anni di tranquilla gestione dell'ordinaria amministrazione perché incombono tuttora sull'Italia questioni di rilievo epocale. Davanti all'impegno necessario per affrontarle, alle opposizioni io non chiedo un voto favorevole; chiedo solo che la loro battaglia politica passi dalla guerra sul numero legale al confronto sui programmi e sulle idee, naturalmente se ne siete capaci.

Indìco, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione nominale con appello della mozione n. 551, presentata I senatori favorevoli alla mozione di sfiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello

Langella,

Comunico che i fogli recanti le firme per la richiesta di *referendum* popolare promosso da un quinto dei componenti del Senato sul testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» sono stati consegnati, su richiesta degli stessi, ai senatori Vito Claudio Crimi, Loredana De Petris e Gian Marco Centinaio, delegati a depositare la richiesta presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 25 maggio 1970 n. 352.

Indìco, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione nominale con appello della mozione Paolo, Centinaio, Bonfrisco e da altri senatori. I senatori favorevoli alla mozione di sfiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

c'è una breve casistica: prima al senatore Gasparri e, in un'altra occasione, al senatore Casson era stato consentito di rivotare, avendo commesso un errore materiale. Penso che la volontà soggettiva di un senatore valga più di eventuali *querelle* e di quanti passi abbia fatto o non abbia fatto una persona. Naturalmente, mi rimetto alla Presidenza. In ogni caso, se

sono i Segretari a decidere su quanto hanno registrato.

pronuncia il voto, l'esito è già acquisito. Far fare un giro ulteriore o, peggio ancora, farglielo fare in retromarcia: due precedenti, due errori, non fanno una cosa giusta.